la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

che, ad ora, non sono ancora giunti in visione ai Gruppi parlamentari. Quindi, non sappiamo esattamente a quale stadio essi siano giunti. È ovvio che ci auguravamo

le chiediamo la garanzia di intervenire affinché il Governo e i relatori procedano al più presto nel metterci nelle condizioni di esaminare i nuovi emendamenti, valutandone nel corso dei lavori anche l'entità, soprattutto avendo riguardo a tempi congrui

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 giunge in Aula dopo una lunga istruttoria nelle Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente. Le modifiche adottate nel corso dell'esame nelle Commissioni hanno ampliato il contenuto del provvedimento, apportando notevoli migliorie al testo, tese soprattutto a prevedere l'introduzione di semplificazioni per le imprese e garantire maggiori tutele per cittadini, territorio e ambiente. Permettetemi di ringraziare i senatori di maggioranza e di opposizione, con i quali abbiamo portato avanti un confronto costruttivo che ha permesso al decreto-legge di giungere in Aula quest'oggi. altresì, doveroso rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici delle Commissioni riunite 8a e 13a per il prezioso supporto che hanno fornito nel corso di queste complesse giornate, in particolare ai dottori Marci e Cavallucci. Venendo ai contenuti, il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; consta di trenta articoli, cui però si aggiungono sei nuovi articoli introdotti nel corso dell'esame nelle Commissioni, suddivisi in tre capi. Il capo I reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area etnea. Il capo III reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017. L'articolo 1, oggetto di diverse modifiche che dettaglierò in seguito, reca numerose innovazioni al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione, recependo alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione pubblica svolta in autunno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dall'8a Commissione, e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. In particolare, il comma 1 reintroduce il regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro centottanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica; autorizza le stazioni appaltanti ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti; prevede che per i lavori pubblici sopra soglia il progetto di fattibilità sia sempre preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali, mentre sotto soglia è facoltà della stazione appaltante richiederne la redazione. Con due modifiche approvate dalle Commissioni riunite (emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.40 (testo 2)) è stato previsto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica debba individuare, tra più soluzioni, quella che presenta - oltre al miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività anche il minor consumo di suolo possibile e che lo studio di fattibilità sia redatto sulla base, tra l'altro, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse. Le Commissioni riunite hanno poi soppresso il periodo introdotto dal decreto-legge all'articolo 24 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione, circoscrivendo, inoltre, con l'approvazione dell'emendamento 1.98, la disciplina dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie Il decreto, con la lettera *b)*, introduce la possibilità che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possano essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici, condizionando però tale possibilità al fatto che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. Anche la disciplina del calcolo del valore stimato degli appalti aggiudicati per lotti distinti è modificata, al fine di prevedere che, in tali casi, sia computato il valore stimato complessivo della totalità dei lotti. Si provvede a estendere la previsione dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture (lettera *e)*, numero 3)). Si modifica, inoltre, la disciplina dei contratti sotto soglia (lettera *f)*), sulla quale le Commissioni riunite sono intervenute con ulteriori modifiche, in particolare prevedendo, per gli affidamenti tra i 40.000 e 150.000 euro (per i

Il decreto-legge prevede poi che le stazioni appaltanti possano sempre decidere, a condizione che sia previsto nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara, che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Le Commissioni riunite hanno chiarito che le stazioni appaltanti che si avvalgano di tale facoltà debbono procedere alla verifica suddetta prima dell'aggiudicazione definitiva. rende inoltre facoltativo per i Comuni non capoluogo di Provincia il ricorso a centrali di committenza, a soggetti aggregatori, a unioni di Comuni o alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane o gli Enti di area vasta, autorizzandoli a procedere direttamente e autonomamente Le Commissioni riunite, mediante l'approvazione dell'emendamento 1.233 (testo 2), hanno poi previsto l'inserimento degli archeologi tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il provvedimento, alla lettera *h),* stabilisce la modifica dei requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi, prevedendo che i consorzi stabili eseguano la prestazione con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto. In caso di appalto integrato, il decreto prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del regolamento di attuazione. Tali requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono invece documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva, ove tali requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione. Si prevede inoltre alla lettera *m)* che, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo nazionale delle commissioni giudicatrici, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle competenze connesse. La successiva lettera *n)* modifica la disciplina dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara. Le Commissioni riunite hanno previsto la soppressione della possibilità di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara nel caso in cui la stazione appaltante possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Le Commissioni hanno altresì modificato l'articolo 83 del codice, in materia di criteri di selezione, prevedendo che i requisiti generali e speciali di cui all'articolo in questione debbano essere posseduti dai concorrenti fino alla conclusione della procedura di gara. Il decreto, alla lettera *p)*, provvede inoltre a chiarire che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio. Gli organismi che rilasciano le SOA svolgono funzioni di natura pubblicistica. Il periodo di attività documentabile è esteso da dieci a quindici anni, al fine di tenere conto della crisi economica che ha determinato l'impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente. Le Commissioni riunite hanno stabilito che, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale, nonché per i subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Il decreto-legge, alla lettera *s)*, ha poi apportato alcune modifiche alla disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto prevedendo, tra l'altro, che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo. Sul punto dei criteri di aggiudicazione, le Commissioni riunite hanno previsto la reintroduzione del tetto del 30 per cento per il punteggio economico ai fini dell'individuazione del rapporto qualità/prezzo, di cui il decreto-legge ha invece sancito l'eliminazione. Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite prevede poi che, nell'offerta economica, devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'operatore economico e che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, Con le disposizioni di cui alla lettera *t)* si provvede, inoltre, a disciplinare le modalità per il calcolo della soglia di anomalia, sostituendo i cinque metodi alternativi finora previsti dal codice con un unico sistema di calcolo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili. Con riferimento alla disciplina del subappalto, le Commissioni riunite hanno previsto che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture (mentre il decreto-legge aveva portato tale percentuale dal 30 al 50 per cento), e hanno previsto la reintroduzione del divieto di affidare il subappalto a chi abbia già partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, del quale il decreto-legge aveva disposto invece l'eliminazione. Restano ferme l'eliminazione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta e l'estensione del pagamento diretto a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore. Le Commissioni riunite hanno inoltre riportato l'incentivo del 2 per cento alle finalità originariamente previste dal codice dei contratti pubblici, eliminando l'incentivo per le attività di progettazione reintrodotto dal decreto-legge. È prevista poi la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale le concessioni già in essere si adeguano all'obbligo di affidare l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica. Si dispone altresì l'ampliamento del novero dei soggetti che possono presentare alle stazioni appaltanti proposte di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, includendovi gli investitori istituzionali. La successiva lettera *gg)* prevede l'eliminazione dell'albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Si demanda la disciplina della qualificazione del contraente generale al regolamento di attuazione, eliminando la previsione per cui l'attestazione del possesso dei requisiti dello stesso avveniva mediante SOA, e prevedendo l'istituzione del sistema di qualificazione del contraente generale, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La lettera *mm)*, numero 6, proroga ulteriormente e amplia l'ambito di applicazione della disposizione transitoria che consente ai concessionari autostradali di avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal concedente stesso, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Ai sensi del comma 3, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice la gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite prevede che, in caso di affidamento diretto, le modifiche apportate dal decreto-legge in esame al codice dei contratti pubblici trovino applicazione qualora, alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, non sia stata ancora avviata la progettazione dell'opera. Le Commissioni riunite hanno inoltre posticipato i termini per l'inizio dell'esecuzione dei lavori per i Comuni beneficiari dei contributi previsti dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici ed edifici comunali che abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti ma non abbiano ancora avviato l'esecuzione dei lavori. I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo. L'articolo 2 reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi, volte a eliminare problemi di coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e la legge fallimentare e a rafforzare il *favor* verso l'impresa momentaneamente in difficoltà, che ha già caratterizzato i recenti interventi in materia di diritto fallimentare. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi infrastrutturali in zone sismiche. In primo luogo, esso apporta una serie di modifiche - volte a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici all'articolo 65 del testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, nonché all'articolo 67, in materia di collaudo statico. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite prevedono che il Ministero delle infrastrutture possa autorizzare laboratori diversi da quelli elencati nell'articolo 59 del testo unico dell'edilizia a effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; dispongono che alcune comunicazioni tra costruttori e sportello unico avvengano tramite posta elettronica certificata e, infine, introducono un termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture deve definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza, nonché delle varianti di carattere sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. L'ultimo articolo di cui sono relatore, il 4, prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più commissari straordinari. I commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche. I commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Essi operano in raccordo anche con Investitalia, la struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, la cui istituzione è prevista dalla legge di bilancio per il 2019. Il comma 6 prevede la nomina di un commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Il comma 7 dichiara conclusi i programmi infrastrutturali «6000 campanili» e «Nuovi progetti di intervento». Le economie risultanti sono assegnate a un nuovo programma di interventi infrastrutturali per i piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. I commi da 8 a 12 disciplinano la realizzazione e il completamento delle opere nelle aree delle Regioni Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, a seguito della cessazione della gestione commissariale. In particolare, alla Regione Campania è affidato il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. L'attuazione degli interventi di completamento sarà vagliato da un apposito comitato di vigilanza, istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Le Commissioni riunite hanno esteso ai contributi, da attribuire ai Comuni per l'anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio per il 2018, le procedure di attribuzione previste per gli analoghi contributi stanziati dalla legge di bilancio per Con riferimento ai contributi ai Comuni previsti dalla legge di stabilità per il 2018, le Commissioni riunite hanno poi previsto che, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, il Ministero dell'interno non proceda al recupero del contributo nei casi in cui il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal Comune. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini previsti, le attività preliminari all'affidamento dei lavori

gli Uffici, sia del Senato che ministeriali. Rivolgo poi un particolare ringraziamento al vice ministro Rixi per il supporto tecnico e politico profuso in questi giorni e anche al ministro Toninelli, nonché ai sottosegretari Crimi e Santangelo. Nel corso della XVIII legislatura è stata posta in essere una serie di provvedimenti legislativi di intervento in favore dei territori del Paese interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni.

circa di queste risorse (ovvero 700 milioni di euro) è stato assegnato nell'anno 2019, mentre per l'esercizio 2020 sono stati concessi circa 238 milioni di euro, pari a circa il 18 per cento del totale delle risorse stanziate. Per l'esercizio 2018 sono state approntate nuove risorse per circa 185 milioni di euro, pari al 14 per cento del totale di risorse previste nel periodo 2018-2023. Infine, nel triennio 2001-2023 sono stati stanziati circa 220 milioni di euro complessivi, con un'assegnazione di risorse man mano decrescente all'avvicinarsi dell'anno terminale del periodo considerato. Nel complesso, le nuove risorse stanziate ammontano a circa 1,35 miliardi per il periodo 2018-2023. In ultimo occorre segnalare che, con la legge di bilancio 2019, sono stati stanziati fondi per circa 360 milioni in favore non di specifici eventi sismici, ma più in generale per emergenze e calamità nazionali.

reca norme in materia di rigenerazione urbana; in particolare, esso prevede che le Regioni e le Province autonome debbano adottare deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sugli *standard* urbanistici, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un aspetto complessivo e unitario, o di specifiche aree territoriali. Ciò al fine di orientare i Comuni nella definizione dei limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati. L'articolo prevede inoltre che, in ogni caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei Comuni della Regione Molise e dell'area etnea indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, contenute nel capo II, articoli da 6 a 20, in via generale dispongono la nomina, in ciascuna delle due aree geografiche,

anche alla riparazione e alla ricostruzione degli immobili privati e pubblici. All'articolo 18 sono state apportate alcune modifiche in materia di struttura dei commissari, prevedendo che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del commissario siano esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura, che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione; che la struttura cessi non alla data di scadenza dell'incarico del commissario (come previsto dal decreto-legge), bensì alla data di scadenza della gestione straordinaria, prevista per il 31 dicembre 2021; che alle spese di funzionamento delle strutture commissariali diverse da quelle indicate nei commi precedenti dell'articolo 18 si provvede nel limite massimo di euro 45.000 per euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021. Le Commissioni riunite hanno previsto l'inserimento all'articolo 7, tra le suddette funzioni, degli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati, nonché il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici. È stato inoltre previsto

l'adozione dei medesimi strumenti. I commissari, infine, sono stati autorizzati ad avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, di Invitalia.

per il quinquennio 2019-2023, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due commissari straordinari, secondo la ripartizione indicata nel provvedimento. Con particolare riferimento alla ricostruzione privata, le disposizioni del decreto-legge prevedono innanzitutto la concessione di contributi per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati distrutti o danneggiati, secondo priorità stabilite dai commissari sulla base dell'entità del danno subito. Esse specificano le tipologie di intervento, di danno e di immobili ammissibili al finanziamento, che può arrivare a coprire il 100 per cento individuando i soggetti beneficiari e disciplinando la procedura per la richiesta e la concessione di contributo; questo agli articoli 9, 10 e 12.

Le Commissioni riunite hanno esteso il divieto di concessione dei contributi, già previsto dal decreto-legge nel caso di immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, ai casi in cui il provvedimento di demolizione o ripristino sia stato impartito

da parte dell'impresa affidataria dei lavori, di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento. Le Commissioni riunite hanno previsto che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica, i commissari sono autorizzati a provvedere direttamente agli interventi per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore e che i commissari acquisiscano i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita conferenza di servizi ai fini della valutazione dei progetti presentati dai soggetti attuatori. Le Commissioni riunite hanno stabilito che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati possano essere affidati dai privati a soggetti che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e che non si trovino in condizioni ostative al rilascio del DURC. Esse hanno inoltre introdotto l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro. Sopra i 40.000 euro resta la procedura negoziata, previa consultazione di dieci soggetti (specificando che debbono essere non genericamente dei professionisti, ma soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici), ma viene eliminato il ricorso al criterio del minor prezzo. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Le Commissioni riunite hanno raddoppiato il contributo straordinario a favore del Comune dell'Aquila, prevedendo non solo 10 milioni per il 2019, ma anche per il 2020 *(Applausi dai Gruppi M5S e 2018 al 31 dicembre 2019 il termine fino al quale le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia sono esentate esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione; amministrazione; - riconosciuto al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle loro attività nel limite complessivo di 80.000 euro per il 2019 e di 80.000 euro per il 2020; euro per il 2020; - specificato che, nel caso in cui i soggetti assunti dai Comuni per gli Uffici speciali per la ricostruzione siano professionisti, è necessaria una dichiarazione di non iscrizione, o avvenuta sospensione, dall'elenco speciale dei professionisti ai quali possono essere conferiti incarichi di

hanno: - introdotto l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro. esecutivo; - previsto che le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, non solo per gli immobili privati che risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", come previsto dal decreto-legge, ma anche "E", limitatamente al livello operativo L4; - consentito - nei comuni che presentano più del 50% di edifici dichiarati inagibili con esito "E" e previa autorizzazione comunale

Infine, si ricorda che le Commissioni riunite hanno previsto l'istituzione di due fondi finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, al fine di assicurare la più ampia tutela a favore rispettivamente dei minori, nei servizi educativi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché dei soggetti ospitati nelle strutture suddette. *(Applausi

nonostante alcune delle modifiche al codice degli appalti siano conseguenti, come sapete, alla procedura d'infrazione che è arrivata dalla Commissione europea,

consideriamo molto negativamente parti rilevanti della proposta che avete fornito con questo decreto-legge. Sono per noi più che evidenti, infatti, le mancate risposte alle varie problematiche emerse sia nella lunghissima indagine conoscitiva come Commissione di merito, sia nelle audizioni svolte. Credo che non si siano mai visti provvedimenti che hanno ricevuto la contrarietà di un così elevato numero di soggetti interessati, protagonisti in questo settore. In pratica è stata chiara a tutti - a noi *in primis* - la duplice volontà, da una parte, di tacitare l'Autorità nazionale anticorruzione, emarginando e comprimendo il principio di legalità, e, dall'altra, di ritornare al vecchio sistema del prezzo più basso,

Siamo convinti che il moltiplicarsi dell'instabilità delle regole, il continuo cambiamento delle norme, proprio quando il codice degli appalti ormai stava entrando in vigore e producendo risultati

assolutamente condiviso: l'abolizione delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, l'ANAC; crediamo che il regolamento governativo che dovrà essere emanato non avrà la stessa valenza culturale che avevano le linee guida; la conferma negativa del limite di 150.000 euro come soglia massima finora prevista per procedure negoziate; il ritorno al meccanismo del prezzo più basso, peraltro integrato con un calcolo astruso

l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica solo agli affidamenti di importo superiore alle soglie previste dall'Unione europea, e la moltiplicazione delle centrali di committenza, Lo stesso dicasi per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese che partecipano alla stessa gara - ciò potrebbe favorire i famosi cartelli - e la reintroduzione dei commissari governativi straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti addirittura con possibilità di deroga delle norme in vigore. Ho citato solo alcuni aspetti sui quali si è manifestata la nostra contrarietà. Recependo anche le sollecitazioni dei nostri tantissimi amministratori del territorio, abbiamo partecipato con spirito costruttivo alla valutazione

Tra le proposte da noi presentate, consideriamo di rilievo quella che è stata approvata. Mi riferisco a quella del collega Mirabelli relativamente all'appalto integrato e, in particolare, alla soppressione della norma che, come sapete, prevedeva la possibilità per gli affidatari di concessione di lavori pubblici di essere anche affidatari dei progetti posti a gara. Delle nostre proposte che sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea ne cito alcune. Noi chiediamo, per esempio, di ripristinare la soglia dei 40.000 euro oltre la quale applicare agli affidamenti la procedura negoziata. Con la legge di bilancio è stata elevata a 150.000 euro. Relativamente alla verifica dei requisiti, dopo l'analisi delle offerte, chiediamo il ripristino delle medesime sull'aggiudicatario da parte delle stazioni appaltanti che abbiamo fatto ricorso alla procedura negoziale. Per quanto riguarda il subappalto, chiediamo di non consentire a chi ha partecipato alla gara senza aggiudicarsela di poter comunque svolgere i lavori come subappaltatore. È evidente che questa proposta negativa, a nostro modo di vedere, accordi tra le imprese durante le gare. Nel merito delle offerte anomale, proponiamo di eliminare i nuovi criteri di calcolo, che di fatto

Sui criteri di aggiudicazione degli appalti, visto che avete tolto la percentuale del 30 per cento per il punteggio economico per le offerte economicamente più vantaggiose, chiediamo di evitare che il punteggio sul prezzo influenzi in maniera preponderante tutte le altre caratteristiche. Per qualificare le stazioni appaltanti abbiamo degli emendamenti che mirano a ridurne il numero, anche concedendo la possibilità ai Comuni non capoluogo di attivarle esclusivamente in presenza di personale che sia adeguatamente formato. Negli anni infatti, abbiamo notato, che questo era uno dei problemi soprattutto per i Comuni più piccoli. Sui controlli, sull'esecuzione e sul collaudo, proponiamo il ripristino delle figure del direttore dei lavori e del collaudo pubblico nel *general contractor*, che non abbiamo più trovato nella vostra proposta. Sui commissari straordinari per le opere prioritarie, come peraltro già osservato nella cosiddetta legge obiettivo del passato, chiediamo di stabilire delle procedure accelerate e semplificate proprio per le grandi opere che più possono mettere a rischio, se mal progettate o mal realizzate, l'esito di questi affidamenti. Di assoluto rilievo è anche la nostra proposta - che è stata approvata, peraltro - del collega Margiotta relativamente alla necessità che i commissari provvedano ad assicurare la ricostruzione attraverso specifici piani di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati e non soltanto con piani di trasformazione e delocalizzazione urbana.

che gli edifici privati distrutti o danneggiati siano riparati o ricostruiti garantendo agli aventi diritto la copertura del 100 per cento del danno subito. In relazione al sisma in Abruzzo del 2009 e a quello dell'Italia centrale del 2016, come peraltro chiesto anche dalle Regioni interessate, chiediamo: di incrementare il personale per gli uffici speciali per la ricostruzione; di concedere ulteriori semplificazioni; un maggiore incremento delle risorse rispetto a quelle ricordate

Sul crollo del ponte Morandi, chiediamo: l'incremento delle risorse per il ristoro dei danni subiti dai cittadini nelle zone di cantiere; il ricalcolo dei tempi per valutare la riduzione del fatturato delle imprese per avere ristoro nonché il rimborso delle maggiori spese subite per i trasporti anche per imprese e liberi professionisti. Chiudo su Radio Radicale.

Spegnere una voca così dettagliata, molto seguita ed unica nel suo genere per costanza ed approfondimenti diretti, sarebbe un pericolo per tutti coloro che tengono alla conoscenza ed alla libertà, principi per i quali - come è noto - molti italiani prima di noi hanno concesso la propria vita per ottenerle.

possa condividerle, per migliorare un provvedimento che - ripeto - anche se in gran parte corretto, così come è non ci soddisfa appieno. Era

evidenzia un'urgenza, quella di scegliere e poi adeguatamente dar corso ad opere infrastrutturali importanti per il nostro Paese; evidenzia anche l'urgenza di intervenire sulle nostre città contro il degrado urbano, urbano, nonché di intervenire per superare una volta per tutte lo stato a volte di abbandono delle aree colpite dal sisma e di quelle legate al disastro vergognoso di Genova. C'è un «però», perché ormai ci siamo abituati in questo anno di Governo-non Governo di questa maggioranza ad avere dei provvedimenti in cui il titolo, o la sintesi comunicativa del titolo, racconta esattamente l'opposto del contenuto. Si potrebbe fare qui una lunga serie di nomi: basti pensare al decreto dignità e a quello che invece ha comportato; era il decreto-legge che doveva abolire in un colpo solo la povertà nel nostro Paese,

ha voluto chiamare sblocca cantieri. In realtà, dimostreremo nel corso del dibattito di questa giornata e delle votazioni di domani con la presentazione degli emendamenti che questo è un decreto blocca cantieri. cantieri. Colleghi, durante le settimane di lavoro e le giornate di audizioni abbiamo potuto vedere plasticamente come questo provvedimento scontenti tutti: dall'ANCE, cioè i costruttori, alle associazioni ambientaliste, da Confindustria ai sindacati, dall'ANAC alla Corte dei conti.

È un provvedimento che cerca - ed è questo il nodo politico - di superare l'incapacità politica di scelta di questo Governo, e in particolare del ministro Toninelli, attraverso una modifica del codice dei contratti. Ma non è con una modifica delle procedure che si supplisce all'incapacità politica di governare e di decidere. Infatti, colleghi, se c'è bisogno di un commissario

perché commissariando Toninelli probabilmente opere fondamentali, anche piccole, di ordinaria manutenzione, si possono fare senza blaterare solamente come sta facendo il Ministro da anni. anni. Colleghi, bisogna anche dire che questa modifica del codice degli appalti ingarbuglia il sistema delle decisioni, perché c'è un problema di tempi, c'è un problema di armonizzazioni, ma anche di comunicazione e di organizzazione. Il codice degli appalti lo avete già cambiato quattro volte in pochi mesi. Questo è il quinto cambiamento in pochi mesi di Governo. Lo avete modificato con il cosiddetto decreto semplificazione nel dicembre 2018, lo avete modificato poche settimane dopo con la legge di bilancio, sempre nel dicembre 2018.

Passiamo adesso all'altra questione centrale, cioè la questione delle città e delle periferie. Questa maggioranza parla di periferie, parla, giustamente, di aree degradate,

topografico, ma dal punto di vista sociologico e culturale. Le periferie sono entrate ormai anche nei centri storici e nei centri urbani. Questa è la verità. Pertanto, un vero piano di investimento strutturale per le nostre città è assolutamente necessario perché attraverso lo sviluppo delle nostre città passa il miglioramento della qualità della vita nonché della crescita economica di tutto il Paese.

Si badi bene che nel comma 1 dell'articolo 5 che presentate, definite degli obiettivi audaci e che noi condividiamo fino all'ultima lettera. Dite infatti che bisogna ridurre drasticamente il consumo del suolo, suolo, favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, agevolare la riqualificazione delle aree degradate, agevolare la riqualificazione degli edifici dismessi o in via di dismissione, agevolare la rilocalizzazione, favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica, favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, assicurare l'adeguamento l'adeguamento sismico anche con interventi di demolizione e ricostruzione. Bene, allora continuiamo a leggere l'articolo per capire come si vogliono raggiungere tali fondamentali obiettivi. E poi scopriamo

alla legge di applicazione (risalente al 1968 che definisce le altezze, le volumetrie, le distanze e le densità urbanistiche), a tutte le leve fiscali e via dicendo. Noi proponiamo un intervento organico, in modo tale che - finalmente - nel nostro Paese si possa fare davvero il bene delle città, delle periferie e dei nostri cittadini.

le aree già occupate e dismesse che non sappiamo come rigenerare. Abbandoniamo e creiamo buchi neri nei centri storici e urbani e, poiché non sappiamo cosa farne, costruiamo fuori occupando terreno vergine. Continuiamo con una politica urbanistica espansiva nel momento in cui l'80 per cento degli edifici residenziali del nostro Paese è della peggiore classe energetica (ossia la G).

La regia pubblica deve poi scendere a livello locale, perché il disegno delle città deve passare attraverso la discussione e la partecipazione pubblica, l'indirizzo dei Consigli comunali e - poi - la capacità di coinvolgimento dei privati. in tutto il mondo si fa rigenerazione urbana solamente se c'è la capacità di avere finanziamenti pubblici accanto a quelli privati. Chi dice il contrario non sa ciò di cui parla.

in questo Paese, continuare ad avere la massima attenzione politica e amministrativa solamente nel momento in cui ci sono i fari dell'opinione pubblica. Non è che i problemi di Genova, dopo il disastro, si superano con un colpo di bacchetta magica. Bisogna costantemente seguirli e il Governo deve farlo quotidianamente. Gli emendamenti che abbiamo presentato, in particolare la senatrice Pinotti, vanno nella direzione di supportare le amministrazioni, le imprese, i professionisti e, soprattutto, i cittadini di tutta quell'area. *(Applausi del

Signor Presidente, premesso che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, rileviamo che nel decreto-legge si prevede la moltiplicazione, a discrezione dell'Esecutivo, di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti. Si tratta di un modello molto simile a quello della Protezione civile durante i Governi Berlusconi, addirittura potenziato, che, per l'indeterminatezza delle norme derogatorie della legge ordinaria contenute nel decreto, si pone in grave contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, che richiede che siano rigidamente determinate per legge le sfere di competenza, le specifiche attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari pubblici. Considerato che la moltiplicazione delle figure commissariali e la contestuale previsione di attribuzioni derogatorie delle norme di legge ai commissari nominati discrezionalmente dal Governo si pone in palese contrasto con il principio di legalità e rischia di portare alla costituzione di una vera e propria amministrazione parallela, non regolata dalla legge, priva della necessaria imparzialità e alle dipendenze dirette dell'Esecutivo, una tale nuova organizzazione amministrativa, istituita discrezionalmente dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con la Costituzione italiana che richiede, all'articolo 97, che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, proprio al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

di uno o più commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e attribuisce a tali commissari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, non è chiarito dalla norma se la disposizione in esame operi in deroga alla disciplina vigente in materia di programmazione delle infrastrutture prioritarie, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di ritenere prioritari interventi infrastrutturali non classificati come tali dagli attuali strumenti di programmazione previsti dalla legge. legge; tenuto conto che: l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori; per i pareri relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio degli atti propedeutici all'approvazione del progetto; la genericità della previsione del silenzio-assenso nei casi in cui è prevista l'acquisizione di nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini senza che nel decreto siano specificamente indicati, con idonei riferimenti normativi, i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici i cui termini risultano oggetto di semplificazione, rischia di porre in pericolo interessi di particolare rilievo costituzionale quali quelli della tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'ambiente; un quindicennio di disastrosa applicazione delle norme derivanti dalla cosiddetta legge obiettivo ha mostrato la pericolosità di procedure accelerate e semplificate proprio per le grandi opere, proprio per le grandi opere, che più possono mettere a rischio, se mal progettate, mal realizzate o costruite nel posto sbagliato, la tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. In fondo era proprio questa impostazione che il nuovo codice appalti del 2016 intendeva superare. altresì valutare che, per la figura del commissario straordinario, introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, era previsto almeno che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti dovessero contenere l'indicazione delle principali norme cui si intendeva derogare ed essere motivati, nelle norme del decreto sui commissari straordinari, non solo tale determinazione non è richiesta, ma non è neppure previsto l'obbligo di motivazione delle deroghe. Nel nostro ordinamento costituzionale vige ancora il principio di legalità il tentativo del Governo di aggirarlo, riservandosi la nomina di soggetti che opereranno al di fuori della legge, lascia i cittadini in balia degli atti arbitrari di commissari di diretta nomina politica, senza alcuna garanzia a tutela della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e consegnando all'arbitrio di pochi l'integrità del paesaggio, la salubrità dell'ambiente e la salute dei cittadini.

e dei beni culturali, garantite dall'articolo 9 della nostra Costituzione. A mio avviso, il punto più delicato e di palese

senza avere neanche un elenco delle opere prioritarie. Vorrei ricordare anche che questo decreto-legge è stato approvato, salvo intese, in Consiglio dei ministri, ha vagato per un mese, poi è stato approvato un'altra volta. È evidente che non vi sono le condizioni per l'applicazione e il rispetto del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Per tutti questi motivi preannuncio

ha recentemente stimato in quasi 600 le medie e grandi opere bloccate, per un valore di ben 50 miliardi di euro, che salgono a oltre 100 miliardi, se si calcolano le ricadute sull'intero sistema economico nazionale. luogo, nella Nota di aggiornamento al DEF dell'anno scorso abbiamo ricordato che in Italia tra lo stanziamento delle risorse e l'effettiva consegna dell'opera conclusa è stato stimato che passano in media due anni per lavori di ammontare inferiore a 100.000 euro, si arriva fino a quindici anni per lavori di valore superiore a 100 milioni. Il motivo è semplice e non lo dico io, ma gli esperti del settore: la metà del tempo - sprecato - è da addebitarsi all'eccessiva lentezza burocratica. In questi anni abbiamo speso appena il 4 per cento dei 150 miliardi di euro stanziati per le infrastrutture e solo il 19 per cento dei fondi europei 2014-2020 (e sottolineo che sono passati già cinque dei e, per finire, appena l'1,5 per cento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinato alla dotazione infrastrutturale del nostro territorio Questa è l'eredità di fronte alla quale si trova l'attuale Governo e restare con le mani in mano, come si è già fatto negli anni passati, non era più possibile. Per la prima volta nella storia il Governo ha dato senza chiedere nulla in cambio, anche alle amministrazioni locali. Ricordo che da poco abbiamo stanziato: 11 miliardi di euro per un piano di tutela del fragile del fragile territorio italiano, ribattezzato «proteggi Italia»; 400 milioni a favore dei piccoli Comuni per le opere di messa in sicurezza delle infrastrutture locali e 500 milioni, sempre a beneficio dei Comuni, per opere di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico. Dobbiamo però anche essere in grado di spendere l'ingente massa di risorse stanziate nel corso degli anni dalle varie manovre, risorse incredibilmente rimaste impantanate nelle sabbie mobili della burocrazia. Il Ministero dell'economia ha certificato infatti che, dei 150 miliardi di euro già previsti nel bilancio (stanziati in quindici anni) per gli investimenti pubblici, ben 118 sono immediatamente attivabili. decreto-legge in esame, lo sblocca cantieri, che ha al suo interno i migliori presidi per il corretto funzionamento delle procedure. Ci tengo a sottolineare l'introduzione di una nuova procedura aperta per appalti di lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero 5,2 milioni di euro, procedura che non prevede affatto l'aggiudicazione della commessa con il criterio del massimo ribasso, come erroneamente e strumentalmente qualcuno ha sostenuto. La norma infatti prevede l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, prezzo, ben diverso dal massimo ribasso, con un meccanismo automatico di esclusione delle cosiddette offerte anomale, ovvero quelle offerte così basse che naturalmente non possono garantire una seria esecuzione dell'opera. Il meccanismo è semplice: prevale l'offerta che più si avvicina alla media dei ribassi. L'azione che mettiamo in campo accarezza diverse discipline: il mondo delle rinnovabili, l'ambiente, i beni culturali, il governo del nostro territorio e, appunto, l'edilizia. Si tratta di diverse sfaccettature per un cambiamento che auspichiamo possa essere tangibile in poco tempo. Infatti, nel breve periodo sbloccheremo fino a 300 opere pubbliche, smascherando la propaganda di chi vuole dipingerci come una forza politica ostile alle infrastrutture. Siamo e saremo sempre contro lo sperpero di denaro pubblico, ma siamo anche parte di un Governo che sta rilanciando gli investimenti pubblici, crollati al minimo storico dell'1,9 per cento del PIL nel 2017. Non è complicando la vita burocratica alle piccole imprese che si combatte la corruzione. Nella legge di bilancio abbiamo messo i soldi per far risalire gli investimenti pubblici al 2,1 per cento del PIL già entro fine 2019 e al 2,7 per cento entro il 2021. Non a caso, i dati dei primi due mesi del 2019 ci danno ragione, con una crescita esponenziale dei pagamenti per appalti e bandi di gara nelle Regioni (+89,4 per cento) e nei Comuni (+21,8 È continuando così, come stiamo facendo, che daremo nuova linfa a un settore che rappresenta il perno centrale dell'economia italiana. L'Italia deve ripartire e grazie alle misure messe in campo da questo Governo finalmente riuscirà a farlo in tempi più veloci.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quello che ci accingiamo a discutere ora è un provvedimento fondamentale per la nostra economia. So che spesso si tende a enfatizzare quello che si fa e quindi si ricorre all'espressione che ho usato poc'anzi. In questo caso, tuttavia, ritengo che la mia espressione sia particolarmente appropriata per una serie di considerazioni. Se, uscendo da qui, andassimo a parlare con imprenditori, liberi professionisti, artigiani e chiedessimo loro quali sono, secondo loro, i maggiori problemi che in questo momento abbiamo nel nostro Paese, riceveremmo quasi sempre la stessa risposta e cioè che il problema sono le tasse e la burocrazia. So che a qualcuno potrebbe sembrare che stia parlando per *slogan*, ma così non è: sono convinto che stiamo parlando di punti programmatici da realizzare

che ridurre le tasse è una necessità per il sistema produttivo di questo Paese. Abbiamo sempre aggiunto che non solo questo migliorerebbe il nostro PIL e la nostra forza occupazionale,

Se tornassimo indietro di qualche decennio, al 1982, per la precisione, a quando Ronald Reagan, in applicazione delle politiche economiche di Laffer, ridusse le tasse, e andassimo a verificare quali sono state le conseguenze, accerteremmo che non solo il sistema produttivo statunitense ne ha beneficiato per i quindici-venti anni successivi, ma che anche il sistema fiscale statunitense ne ha beneficiato in egual misura. Non a caso, infatti, per quasi dieci anni consecutivi, dal 1982 al 1990, il gettito per l'erario aumentò tutti gli anni, passando dai circa 600 miliardi di dollari

agli esempi virtuosi europei di quegli Stati che crescono più degli altri o che superano più agevolmente le crisi, troveremmo che in queste realtà c'è sempre un sistema di tassazione fissa, come la *flat tax* che vogliamo introdurre noi, che è comunque a livelli molto bassi. Anche in Italia abbiamo un esempio positivo in tal senso, perché quando fu introdotta la cedolare secca molti dicevano che era una misura che non avremmo potuto per metterci,

quel periodo degli anni Sessanta quando l'Italia cresceva più di chiunque altro, troveremmo che una delle peculiarità del nostro Paese era un livello impositivo più basso di quello di molti altri Stati; non era quindi un caso

anche la nostra produttività si è allineata; ugualmente, non è stato un caso che quando il nostro livello impositivo è diventato più alto di quello degli altri Paesi, la nostra produttività e la nostra competitività sono crollate e ci siamo ritrovati ad essere non solo fanalino di coda di coda in Europa, con livelli di crescita o decrescita sempre peggiori rispetto a tutti gli altri, ma anche un pessimo esempio a livello mondiale. Per in un momento di difficoltà come quello attuale, in presenza di una economia debole come la nostra, un provvedimento che risolve uno di questi due problemi, cioè quello della possibilità di far partire i lavori, quindi di semplificare la burocrazia, è fondamentale. Il provvedimento in esame reca misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in attesa di poter abbassare le tasse (altro punto programmatico del nostro partito), è sicuramente la migliore soluzione che potremmo proporre al nostro Paese in un momento di difficoltà

senza considerare che la guerra dei dazi in atto e le altre criticità internazionali potrebbero pregiudicare ulteriormente uno scenario che già positivo non è. Pertanto, far partire i lavori, far partire quello che potrebbe diventare, anzi che sicuramente diventerà il più grande cantiere d'Europa è una risposta rapida, efficace e una delle poche che possiamo permetterci, vista la situazione dei nostri conti pubblici. Ho accennato a quello che sarà il più grande cantiere d'Europa, così entro anche nel dettaglio di alcune misure che abbiamo previsto nel decreto-legge in conversione, e cioè quelle a favore delle popolazioni terremotate. Sappiamo bene che, purtroppo, un'impostazione eccessivamente farraginosa e burocratica della ricostruzione ha impedito fino ad ora la partenza dei cantieri.

potrà rappresentare una risposta non solo a quelle persone che hanno solo una richiesta tra le proprie priorità, cioè rientrare nelle proprie case, ma anche una risposta positiva in termini di occupazione e di PIL. facendo di nuovo riferimento agli insegnamenti della storia, è dimostrato che far partire la realizzazione di opere (poco importa se pubbliche o private) non fa altro che risollevare l'economia in difficoltà. Ce l'ha insegnato il piano Marshall, che, dopo la Seconda guerra mondiale e con una situazione compromessa dal conflitto, non ha fatto degenerare le conseguenze dello stesso, ma ha anzi permesso una ripresa dell'economia. Leggo testualmente la dichiarazione di Marshall quando ha presentato il piano, adottato appunto per evitare quello che definiva «Un gravissimo deterioramento delle condizioni politiche, economiche e sociali», proprio perché - come dicevo prima tutte le misure che favoriscono l'occupazione, tutte le misure che favoriscono il lavoro e tutte le misure che favoriscono l'economia non possono che, inevitabilmente, favorire tutta la popolazione le misure che ci apprestiamo ad approvare ora avranno conseguenze positive su tutti gli aspetti della nostra vita.

23, comma 1, lettera *a)*, che prevede la possibilità per i Comuni di concordare con gli uffici speciali per la ricostruzione il trasferimento delle istruttorie agli uffici tecnici comunali delle case che hanno avuto esito E con livello operativo L4. Per chi non è un tecnico, mi riferisco

Questa misura non solo agevolerà molto la ricostruzione dei paesi distrutti, perché evidentemente si rivolge a quelli, ma consentirà finalmente

signor Presidente. Più volte in quest'Aula si è criticato il fatto che già oggi ci vogliono troppi mesi per l'approvazione dei progetti. Consentire ai Comuni di gestire le istruttorie su queste pratiche non potrà che agevolare il tutto. Ci sono molte altre previsioni, sia a favore delle popolazioni terremotate che a favore di chi è in una situazione di debolezza e difficoltà (come ad esempio le telecamere negli asili nido e nelle case di cura); sono certo che i miei colleghi saranno più esaustivi con riferimento a questi provvedimenti. *(Applausi

quella degli appalti pubblici è una materia complessa e delicata, perché in essa da sempre si annida il serio rischio della corruzione e della concussione e perché è il tramite attraverso cui i comitati d'affari e la criminalità si legano alla politica. Lo sblocco, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure in questo settore, spacciate come un taglio alla burocrazia, sono state più volte all'origine di provvedimenti che, invece di favorire aziende e lavoratori, hanno solo aumentato il lavoro di magistrati e Forze dell'ordine. Le modifiche che stiamo discutendo costituiscono il ritorno a un vecchio armamentario, che speravo essere stato superato con l'introduzione del nuovo codice degli appalti. Questo decreto-legge ha ben poco a che vedere con lo scopo di sbloccare i cantieri, ma sembra più riguardare in generale uno sblocca corruzione, un allentamento delle regole di trasparenza e vigilanza, una sottovalutazione del rigore necessario per le autorizzazioni, così diminuendo la tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Non ho molto tempo a disposizione per evidenziare tutti i passaggi critici, ma vorrei sottolineare negativamente almeno il ritorno, fino al 2021, dell'appalto integrato, il vecchio appalto concorso, ovvero la progettazione ed esecuzione dei lavori da parte dello stesso soggetto. La progettazione indipendente da chi deve realizzare l'evento è stato uno dei capisaldi del nuovo codice degli appalti e aveva lo scopo di incrementare la qualità dei progetti e la ricerca di soluzioni tecnologiche che che al meglio potessero inserire le opere nel contesto ambientale, territoriale e urbano. Il ritorno al vecchio regime viene inoltre completato dalla riesumazione - ahimè - dei commissari straordinari. A tal proposito, considerata l'ampiezza dei poteri di deroga riconosciuti ai commissari, sarebbe stato opportuno prevedere l'obbligo almeno di motivazione delle deroghe. Per questo ho presentato un emendamento, che mi auguro possa essere accolto. Un ritorno al passato è generato anche dalle proroghe sulla quota di lavori da mettere a gara per le concessioni, dall'aumento del subappalto, dagli allenamenti dei controlli e della soglia dei lavori a trattativa privata, dalla destrutturazione delle procedure autorizzative in materia di infrastrutture strategiche, soluzioni già sperimentate in passato, che non hanno assolutamente incrementato i lavori, ma solo la scarsa qualità delle opere pubbliche, talune rimaste incompiute e inoltre un aumento ingiustificato dei costi, oltre che, come ho già detto, gravi episodi di corruzione e di concussione. Cari colleghi della maggioranza, a poco serve lanciare messaggi di rigore con una mano, se con l'altra si alza a dismisura la soglia per gli affidamenti diretti di lavori senza gara, se ritorna il criterio del prezzo più basso per lavori di milioni di euro, se si reintroduce la libertà di subappalto, se si cancellano le linee guida dell'anticorruzione. Ai colleghi 5 Stelle dico: non eravate quelli della legalità, dell'onestà, della trasparenza? Questo provvedimento, come altri che avete votato in quest'ultimo anno, va - sappiatelo, ma lo sapete - nella direzione opposta. Gli elettori se ne sono accorti,

Signor Presidente, colleghi senatori, dopo oltre un anno dall'avvio della legislatura sembra che finalmente questo Governo si sia accorto che rimandare, analizzare, ripensare e infine tentare di cancellare ogni opera che possa creare lavoro, crescita e sviluppo non sia esattamente quello di cui il Paese ha bisogno. A noi, in verità, pareva che non fosse così difficile capire che alle persone interessa legittimamente che si creino le condizioni per consentire di fare impresa, di dare lavoro, di lavorare, di spostarsi velocemente e in modo sostenibile tra le nostre città e verso l'Europa e il mondo. Per questo non abbiamo mai smesso di sostenere le idee giuste, di lavorare a progetti che consentano di ridurre le tasse, di rendere lo Stato più efficiente, di migliorare la scuola e l'università, di proporre investimenti in ricerca e sviluppo, di utilizzare le opportunità che arrivano dall'Europa, di portare a termine i tanti progetti infrastrutturali che possono rendere il Paese più competitivo. Ora pare che almeno sul fronte dei lavori pubblici il Governo si sia accorto di quanto sia necessario non rimandare ma agire, non analizzare e ripensare ma portare a termine. Prendere atto del presunto risveglio del Governo porta però con sé almeno due considerazioni. La prima è che se è necessario un intervento che consenta di avviare o riavviare i cantieri, allora tutte le premesse di metodo che questo Governo si era dato fino a qui, ovvero che le opere dal TAP al TAV non dovessero essere portate a termine, cadono. Erano premesse sbagliate ed è tempo che il Governo lo ammetta esplicitamente. La seconda considerazione che il decreto-legge che ci accingiamo a convertire induce naturalmente a fare è che, nonostante il tentativo ancora una volta, non basta usare una formula linguistica per riuscire a fare le cose per bene. La formula apparentemente accattivante dello sblocca cantieri, infatti, non è sufficiente perché i cantieri si sblocchino, perché si passi dal dire al fare. Naturalmente sappiamo benissimo perché si è scelta questa formula apparentemente evocativa, «sblocca cantieri»: l'idea è di far credere ai cittadini - o forse dovremmo dire agli elettori che anche un Governo che sta in piedi grazie a un ben orchestrato disaccordo permanente e che più che agire tende a tirare a campare possa fare qualcosa per lo sviluppo, la crescita e lo sblocco di quello che nel Paese c'è da sbloccare. Purtroppo, non è così: è così: ancora una volta, il decreto-legge, lungamente meditato dal Governo, con tempi biblici tra l'annuncio e la pubblicazione, non ha contenuti all'altezza nemmeno della formula con la quale è stato sintetizzato, la quale va dunque da subito ridefinita, perché qui siamo certamente davanti ad un intervento che non sblocca i cantieri. I decreti e i provvedimenti attuativi presenti nel testo si sprecano e quindi trascorreranno ancora mesi prima che il quadro, variamente ipotizzato, possa trovare un'implementazione concreta. Inoltre, ancora peggio sono le molteplici criticità di merito contenute nel testo e rispetto alle quali la maggioranza ha deciso di non intervenire, non solo quando le critiche costruttive sono arrivate dall'opposizione, ma anche - e questo è ancor più grave - quando sono giunte dalle diverse realtà audite, dal Paese dunque, che ancora una volta questo Governo intende non ascoltare. Si propone così uno sblocca cantieri che, anche se fosse stato ben congegnato, sarebbe stato un pannicello caldo. Non si guarda però a chi crea lavoro e a chi lavora, non si incentiva a dovere il riuso edilizio, non si dicono finalmente parole chiare sulla prosecuzione di opere fondamentali come il TAV, il Terzo valico o l'Autostrada 33. È tempo che questo Governo agisca in modo fattivo e incisivo, non solo attraverso mere dissimulazioni lessicali. Il Paese ha bisogno di crescere e guardare al futuro. È tempo che questa maggioranza, insieme ai cantieri, sblocchi se stessa e decida se intende lavorare veramente per l'Italia o se non preferisca invece desistere.

il tema di cui discutiamo (contratti pubblici, accelerazione di interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana) insiste sul codice degli appalti, già oggetto di alcuni nostri interventi: nel decreto-legge sulle semplificazioni, con un'elencazione tassativa e non più esemplificativa dei casi d'illecito professionale; nella legge di bilancio, sugli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni statali, centrali e periferiche; sulla messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; sull'individuazione di una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, proprio per la velocizzazione delle attività di progettazione; nel decreto-legge sicurezza, che ha introdotto una nuova fattispecie di procedura negoziata per un periodo limitato e per i lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria; nel decreto-legge su Genova, con l'introduzione di un archivio informatico nazionale per alcune tipologie di opere pubbliche. Questo per dire che il Governo in carica, fin da subito e con ogni provvedimento con cui è stato possibile, ha cercato di porre rimedio alle criticità e ai punti di confusione esistenti nel nuovo codice degli appalti del 2016, perfino aggiornato nel 2017. Lo sblocca cantieri è il risultato di uno studio e di un lavoro solleciti su princìpi fondamentali, per un effettivo intervento in un settore molto delicato, ma determinante, come quello dei contratti pubblici, su cui raramente s'interviene in modo efficace e tempestivo. Una prima novità di questo provvedimento è la reintroduzione del regolamento unico attuativo del codice degli appalti, che disciplinerà i contenuti della progettazione nei tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) e il contenuto minimo del quadro esigenziale che le stazioni appaltanti devono predisporre, snellendo notevolmente le previsioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 23 del codice degli appalti mai attuato. Si introduce una disciplina semplificativa direttamente applicabile per l'affidamento dei contratti che prevedono manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non contemplino la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali di opere o di impianti. quindi di un *modus operandi* semplificato, che consente l'affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, che abbia un contenuto informativo minimo indicato dalla norma stessa, e la possibilità di eseguire lavori senza redigere o approvare il progetto esecutivo. In realtà, non si eliminano i livelli di progettazione, come qualcuno erroneamente sostiene, ma si interviene sulla norma *ex* articolo 23 del codice degli appalti, solo permettendo che l'espletamento della prima fase non sia più condizionato dal contesto, ma unicamente dall'importo del contratto, relativamente ai lavori pubblici sopra o sotto soglia di rilevanza europea. In merito poi all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si allinea la disciplina della partecipazione di gara nelle concessioni di lavori pubblici dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara alla disciplina europea, secondo la quale i concessionari uscenti che abbiano predisposto la progettazione da porre a base di gara hanno diritto di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento delle concessioni dei lavori pubblici. Si snellisce la procedura di affidamento dei lavori sotto soglia permettendo la previa consultazione di soli tre operatori anziché dieci e si amplia l'ambito di applicazione a tutti i lavori di importo fino a 150.000 euro e ovviamente pari o superiori a 40.000 euro. Per gli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea viene previsto l'affidamento tramite ricorso alle procedure aperte con partecipazione quindi di tutti gli operatori economici dotati di qualifiche e caratteristiche adatte all'affidamento di un determinato appalto e con il criterio del minor prezzo. queste modifiche vanno nell'unica direzione di permettere una velocizzazione delle procedure di affidamento nella piena legittimità delle procedure stesse e il fatto che per quelle sotto soglia la stazione appaltante possa prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia garantisce la tutela di possibili situazioni illegittime. Vengono soppressi i commi 2-*bis* e 6-*bis* dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo relativamente al rito superaccelerato che, pur essendo conforme al diritto europeo, presenta il limite dell'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti a una gara d'appalto dei motivi di illegittimità del provvedimento, che sarebbero onerati di impugnare subito, con la compromissione del diritto di difesa, con oneri a carico dell'impresa e senza raggiungere di fatto l'accelerazione delle procedure di affidamento. Pertanto, adesso i vizi relativi alla fase di ammissione alla gara potranno essere fatti valere nelle forme ordinarie. Si dispone, con attenzione anche per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la conclusione dei programmi infrastrutturali, di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 per la realizzazione di opere pubbliche. Nello stesso ambito, si prevede l'assegnazione a un nuovo programma di interventi infrastrutturali per Comuni fino a 3.500 abitanti dalle economie risultanti dai precedenti programmi per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali. Per la rigenerazione urbana si prevede la necessità e non più solo in via facoltativa, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dell'approvazione di disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 relativamente ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati con adeguamento da parte dei Comuni dei propri strumenti urbanistici, introducendo un contenimento del consumo di suolo, una rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, una riqualificazione delle aree urbane degradate, uno sviluppo dell'efficienza energetica e un miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Concludo affermando con sicurezza che questo provvedimento, fortemente voluto dal Governo e sostenuto da questa maggioranza, darà finalmente impulso al sistema produttivo del Paese, costituito dalle imprese italiane che in questo particolare periodo di stagnazione economica hanno bisogno di essere supportate nella loro attività attraverso l'introduzione di misure di semplificazione del quadro amministrativo e normativo. Consentirà un celere utilizzo delle risorse economiche previste per gli interventi infrastrutturali indifferibili, per gli interventi necessari nelle zone sismiche snellendo l'*iter* burocratico, per gli interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità, per gli interventi edilizi di rigenerazione urbana, per i servizi mobili di comunicazione nei territori interessati da gravi emergenze. Tutto ciò si compie nell'unico, esclusivo e predominante interesse dell'Italia e dei cittadini italiani.

in questa legislatura noi abbiamo sempre avuto una posizione non pregiudiziale nei confronti dei provvedimenti presentati dal Governo, comportandoci secondo correttezza e in base al programma, e quindi alla direttrice che ci siamo dati con i nostri elettori di centrodestra. Tanto meno abbiamo avuto un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di questo decreto-legge,

a cui il Vice *Premier* e Ministro dello sviluppo economico si riferiva all'inizio dell'anno corrente, annunciando per quest'anno, appunto, il miracolo economico. Non è il piano Marshall e non lo è anche perché qui davanti a noi in quest'Aula non c'è il generale Marshall; non c'è nemmeno il Ministro delle infrastrutture.

proprio perché lui stesso e questa maggioranza non danno alcun valore a questo provvedimento. Ciò a fronte di un problema che esiste nel Paese. infatti vero, come è stato detto durante le audizioni delle parti sociali, purtroppo tutte critiche nei confronti del provvedimento, che vi sono 150 miliardi di euro di infrastrutture che potrebbero essere realizzate.

6 miliardi, cioè nulla. I 150 miliardi potrebbero essere sì un piano Marshall, ove fossero sbloccati. Saranno sbloccati? L*'iter* di questo provvedimento è emblematico: è stato approvato una prima volta, poi riposto nel cassetto, poi ripresentato, dopo un altro mese, per essere riapprovato con modifiche, quindi presentato in Parlamento e, da un mese, attendiamo di discuterlo in quest'Aula, perché avrebbero dovuto mettersi d'accordo, in campagna elettorale, sulle modifiche da apportare per migliorare il provvedimento e sbloccare davvero i cantieri. Addirittura, la Lega aveva presentato un emendamento in Commissione per imporre chiarezza sulla realizzazione del TAV, dei treni ad alta velocità e quell'emendamento è stato ritirato dalla Commissione e ci giunge voce che sarà presentato sotto forma di palliativo, cioè di ordine il giorno, ossia di nulla, di fuffa. Ma non lo sappiamo ancora, perché gli emendamenti devono ancora essere presentati. Sono passati tre mesi e siamo ancora in attesa della versione che la maggioranza ricamerà nel presentare questo emendamento. Ciò a fronte di 150 miliardi di euro bloccati e che restano bloccati, perché la misura di questo Governo è lo stallo, il blocco. Quanti decreti attuativi avete fatto della manovra economica finanziaria che avrebbe dovuto cambiare le magnifiche sorti di questa legislatura? Ne avete fatti 20 su 345: il 16 per cento, cioè: tutta la grande manovra economica del Governo è bloccata dalla mancanza di decreti attuativi. Ci giunge notizia che alla Camera hanno sospeso le Commissioni sul decreto-legge crescita. Di quest'altro grande binario dello sviluppo, insieme al decreto-legge sblocca cantieri, che è stato fermato alla Camera in attesa che il Governo e la maggioranza si mettessero d'accordo in campagna elettorale,

tale dalla stessa Lega: l'85 per cento dei piemontesi ha votato forze - in gran parte di centrodestra ma anche altre - che sono nettamente favorevoli ai treni ad alta velocità. C'è stato un plebiscito nelle elezioni laddove sei milioni di elettori hanno abbandonato i 5 Stelle. E il Governo cosa ha deciso? Che domani, a fronte di questo plebiscito, non riunirà il Consiglio dei ministri

20.000 persone iscritte e "blindate" che voteranno secondo un certificato non riconosciuto tale dall'Autorità che garantisce la *privacy*, e quindi anche l'informatica.

la fiducia al *lider máximo* Di Maio e in attesa che 20.000 persone decidano - o meglio che Casaleggio decida - il Governo sospende le attività. Per cui oggi il *premier* Conte si è recato dal Capo dello Stato, dopo aver visto i Vice *Premier*, e ha detto a tutti che ha un'agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare che ci impegnerà per il resto della legislatura e che attende il *referendum* della piattaforma Rousseau. Per sapere se la legislatura potrà continuare, 20.000 cittadini decideranno a fronte di 50 milioni di elettori che hanno già deciso domenica scorsa ed è chiaro il loro responso. e a fronte della paralisi che riguarda tutti i provvedimenti, mi sapete dire quante delibere ha fatto il CIPE? A me risulta che il Comitato interministeriale per la programmazione economica sia fermo da mesi e che venga bloccata ogni decisione. Mi sapete dire qualcosa del provvedimento sui risparmiatori truffati dalle banche e sui decreti attuativi, annunciati e strombazzati in campagna elettorale? Oppure sul cosiddetto decreto crescita paralizzato alla Camera? I risparmiatori otterranno mai quello che avete promesso più di un anno fa? anno fa? Questo Governo, quando legifera, lo fa male guardando soltanto ai titoli - e posso dire che sotto il vestito dei titoli non c'è nulla o quasi nulla - e poi viene paralizzato completamente dai decreti attuativi che non sapete scrivere.

di un decreto sblocca-cantieri; ci sarebbe sì bisogno di investimenti nelle infrastrutture; ci sarebbe sì bisogno di semplificazione e sburocratizzazione e per quello che c'è, ancorché la montagna del titolo - sblocca-cantieri - abbia partorito un piccolo topolino,

il quale tutti gli osservatori internazionali hanno mandato anche delegazioni per capire se davvero il Paese di Casaleggio consentirà a Di Maio di poter continuare la legislatura e a noi di sorbirci l'agenda fitta di impegni del *premier* Conte, sottoposta oggi ai due Vice *Premier* prima di recarsi dal Capo dello Stato (tornandosene con cosa?). Entro venerdì dovrete dare una risposta alla Commissione europea in merito al *deficit* e al debito che quest'anno si è accresciuto. Quella risposta chi la scriverà se il Consiglio dei ministri domani non si può riunire perché attende il responso di Casaleggio? Io credo che quella risposta l'abbiano già data gli italiani e noi ci auguriamo che la diano in maniera ancor più convinta e libera alle prossime, imminenti, elezioni politiche.

perché, come abbiamo detto in Commissione, siamo disponibili a presentare i subemendamenti senza interrompere la discussione in Aula. Chiedo pertanto al Governo almeno di posticipare

non credo sia vera. Che ci sarebbe stata una sola ora di tempo tra la presentazione degli emendamenti agli Uffici e il termine per la presentazione dei subemendamenti è una cosa che a noi non risulta essere stata decisa da nessuna parte con il consenso dei Gruppi. Anzi, si

Non mi pare una richiesta stravagante. Ed è una richiesta alla quale credo che la Presidenza possa accedere.

Una particolare menzione ai relatori, senatrice Faggi e senatore Santillo, per la competenza e la passione messi a disposizione di tutti. *(Applausi dal Sbloccare i cantieri, semplificare le procedure - rese a volte troppo soggettive nell'applicazione del codice appalti - vuol dire fare rialzare la testa all'Italia, farla ripartire. Far ripartire un Paese rimasto bloccato per le politiche miopi degli anni passati. Rigenerare dei vuoti urbani, dare norme chiare e subito applicabili per restituire aree intere alla città, vuol dire rendere più vivibili i nostri territori. Io ho fatto il sindaco, so cosa vuol dire voler fare, saper di dover fare e non riuscire per la troppa burocrazia. Chi si è trovato come me a fare l'amministratore locale o il professionista sa cosa vuol dire trovarsi di fronte ad alcuni articoli del codice degli appalti, nella difficoltà di applicazione, nei dubbi interpretativi dei tecnici comunali, poco incentivati nel trovare soluzioni rispetto alla troppa responsabilizzazione nell'interpretazione delle norme. Questo, insieme ai tagli degli enti locali (solo nell'ultima legge di bilancio sono stati sbloccati finalmente gli avanzi di amministrazione per gli enti virtuosi), ad un blocco totale degli investimenti pubblici locali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. All'interno del provvedimento si rende giustizia a tutti quei Comuni che si vedevano esclusi nella allocazione di risorse dai bandi per opere di messa in sicurezza dei territori, che prevedevano criteri assurdi, stabiliti dal passato Governo, con assegnazione dei fondi esclusivamente ai Comuni in dissesto finanziario, creando una vessazione enorme verso quei Comuni che avevano dato corretta prova di buona amministrazione. Rivedere le soglie per l'affidamento dei lavori per poter sveltire le pratiche è fondamentale per accelerare e poter fare affidamenti diretti, senza ritenere a prescindere colpevoli amministratori locali, tecnici o imprese. Per la consistenza e diffusione sul nostro territorio, il settore degli appalti pubblici costituisce una leva importante della nostra economia. Se l'intenzione del legislatore con il codice dei contratti pubblici era quello di rendere più razionale la spesa pubblica e più trasparente il processo, nella realtà, si è tradotto in una forte aggregazione della domanda, con un peggioramento dell'accesso al mercato da parte delle medie e piccole imprese, che sono un vanto e un patrimonio da salvaguardare, da aiutare a crescere e non a chiudere,

ma riducendo gli oneri a carico delle imprese, facilitando l'accesso alle nostre piccole e medie imprese e, rendendo chiare le norme per una facile applicazione, evitando che le interpretazioni portino a contenziosi dietro ogni angolo, che fanno rallentare la nostra economia. Il settore delle costruzioni in questi anni ha sofferto molto. Migliaia d'imprese hanno chiuso i battenti per la crisi, migliaia di competenze e posti di lavoro sfumati. Ecco: far ripartire i cantieri vuol dire dare nuova linfa vitale al settore, un settore strategico per la nostra economia. Ecco perché questo provvedimento, insieme al decreto crescita in arrivo, è importante; ecco perché i vincoli imposti dall'Europa dimostrano che questa non conosce il Paese Italia, un Paese come il nostro, fatto di tante piccole e medie imprese, fatto di 8.000 comuni, che basa le sue politiche nel contatto diretto con il cittadino; un Paese che per forza deve rivedere quei vincoli europei che hanno bloccato i nostri investimenti e che noi come legislatori abbiamo il dovere di rivedere. Con questo non si vuol dire che siano meno importanti le grandi opere infrastrutturali di cui abbiamo necessità e che noi riteniamo fondamentali, ma non dobbiamo dimenticare il bisogno e la necessità immediata di manutenzioni ordinarie e straordinarie, alle scuole, alle strade, ai ponti, agli edifici pubblici, che beneficeranno dell'accelerazione delle pratiche e che saranno di conseguenza un beneficio della nostra economia. Per troppo si è stati fermi. Serve ripartire, serve crederci. Questo è un inizio, non certo la soluzione di tutto, ma un buon inizio. Ripartiamo.

non se la merita; mi limiterò quindi a far osservare le incongruenze o le problematiche che gli inserti al vecchio codice dei contratti creano o creeranno.

ad esempio, nel caso dei motivi di esclusione da una gara d'appalto, la seguente situazione: il testo precedente diceva che se un subappaltatore fosse stato condannato per tutta una serie di reati in via definitiva, compresi quelli di tipo associativo

per cinque anni abbiamo detto che era un grande problema la tematica del subappalto. Ebbene, il subappalto ritorna più forte che mai. la vecchia normativa escludeva che chi perdeva in una gara d'appalto potesse partecipare come subappaltatore per chi aveva vinto la gara e questo al fine di evitare i cartelli; adesso questa eventualità è di nuovo ammessa. Il caso Lombardia e gli arresti legati proprio a questo tipo di fattispecie evidentemente non hanno insegnato niente e non hanno fatto neanche giurisprudenza in senso negativo. Un'altra previsione che lascia molto perplessi ed è stata anche sollevata in sede di pregiudiziale è la seguente: la Corte costituzionale ha più volte ribadito che l'utilizzo di un commissario straordinario è una compressione dei diritti costituzionali. Ebbene, la si potrebbe giustificare quando il commissario arriva *ex post*, cioè deve risolvere una situazione che si è incagliata per eccesso di normazione, ma qui viene messo nero su bianco che ci sarà un elenco di opere prioritarie (non ancora presente) per le quali il commissario arriva in anticipo: è un commissariamento preventivo e chiaramente una previsione al di fuori della Costituzione, visto e considerato che per cinque anni abbiamo detto abbiamo detto che la via ordinaria era l'unica che andava perseguita. Improvvisamente questa condizione viene completamente cancellata e addirittura la si ammette in via preventiva. Per non parlare del fatto che il commissario arriva e ha la possibilità di andare in deroga a tutto

a scompaginare le carte sulla rigenerazione urbana e sul disegno di legge sul consumo di suolo che stiamo discutendo e per il quale abbiamo fatto oltre ottanta audizioni in Commissioni riunite ambiente e agricoltura. C'è una frase pericolosissima all'interno di questo contesto, ove si dice che prima le Regioni potevano produrre legislazione su materie di competenza nazionale per quanto riguarda la rigenerazione e l'utilizzo del suolo; adesso non è più una facoltà ma diventa un «fatelo»: le Regioni procedono a farlo. In questo modo, prima ancora di poterlo capire, le Regioni avranno messo mano ai piani regolatori e ai piani di espansione e avranno potenzialmente fatto un disastro contro la normativa nazionale che in questo caso è di competenza dello Stato. Questa è una previsione pericolosissima.

È stato inserito un "pezzettino", una modifica che consente di far partire i lavori per chi ha vinto la gara senza aspettare i tempi dei ricorsi. Sappiamo che c'è un ricorso strumentale al ricorso, però faccio una domanda per la quale non c'è risposta. Supponiamo che uno vinca faccia l'opera, arrivi fino in fondo e che poi uno dei perdenti vinca il ricorso. In questo caso chi mette mano al portafoglio per un eventuale risarcimento? Non è chiaro, mentre la norma dovrebbe prevederlo, perché non ferma il ricorso strumentale, ma apre la porta a ricorsi *ex post*

è già in revisione il vecchio codice dei contratti, per cui una manomissione così pesante non aveva veramente ragione di esistere. Grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Atto Senato in questione è stato concepito al fine di dare il via alla ripresa dei lavori pubblici: cantieri, attività produttive e quant'altro possa rappresentare il «primo motore immobile» dell'inizio e della prosecuzione delle attività che contribuiranno alla crescita economica nel nostro Paese. Il capo I del decreto battezzato «sblocca cantieri» non rappresenta, come molti hanno affermato, la riforma del codice degli appalti, ovvero del decreto legislativo n. 50 del 2016: ha sostanzialmente una funzione propedeutica a quella che sarà la vera e propria riforma del codice degli appalti e che questo Governo ha in programma di realizzare. Le modifiche introdotte hanno come obiettivo prioritario la semplificazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti attraverso il recepimento di alcune delle più significative indicazioni pervenute nell'ambito della procedura di consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formulate direttamente dalle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, le quali, in virtù della loro esperienza quotidiana sul campo, hanno la piena consapevolezza delle criticità insite nell'attuale apparato normativo. Fra le modifiche introdotte al capo I del decreto corre l'obbligo di segnalare: l'intervento in materia di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, che possono essere affidati sulla base del progetto definitivo; la modifica delle soglie per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziale e di quelle relative ai subappalti; l'ampliamento dei casi in cui è possibile procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo e la modifica dei meccanismi di determinazione della soglia di anomalia (che hanno generato nella precedente esperienza difficoltà applicative e rilevanti contenziosi), per concludere con l'introduzione di regole che daranno ai progettisti che collaborano con l'appaltatore maggiori certezze sui pagamenti dei loro compensi. Cari colleghi, consentitemi di focalizzare l'attenzione sugli interventi di riparazione e ricostruzione post-sisma, in particolare nella mia amata terra, la Sicilia, e più precisamente nei nove Comuni colpiti dal sisma cosiddetto di Santo Stefano, del 26 dicembre scorso, cioè Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo e Aci Catena.

cui le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, che hanno disciplinato i primi aiuti urgenti conseguenti all'evento sismico che ha interessato l'area etnea, volti ad arginare lo stato di confusione, smarrimento e incertezza del futuro che ha pervaso la popolazione interessata. Sin dalla prima notte, tutte le famiglie, i cittadini sono stati messi nelle condizioni di dormire sotto un tetto, in strutture ricettive locali, ad eccezione di coloro che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. La macchina degli interventi, quindi, si è messa subito in moto. Tutto quanto fosse di competenza del Governo centrale è stato posto in essere, registrando, purtroppo, la non sempre tempestività nello svolgimento degli interventi di precipua pertinenza degli enti locali, nonché un'informazione pubblica spesso disinformata

e dieci dal sisma che ha interessato la città di Campobasso, si potrà dare ristoro a quei cittadini, Comuni e aziende che da tempo attendono questo momento. Inoltre, sono stati previsti contributi straordinari e interventi vari finalizzati all'accelerazione della fase di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale e dell'Aquila, colpite dal sisma del 2016-2017 e del sisma Ritengo importante precisare che il Governo, che si fa prossimo alle esigenze della popolazione, non può limitarsi allo stanziamento di fondi, per poi, periodicamente, dover rimpinguare le casse di Regioni e Comuni a causa di una mancata oculata programmazione di attività di ricostruzione. Ecco perché vi è la necessità di richiedere una proroga dei tempi di realizzazione dei lavori (e, a mio avviso, anche di ristrutturazione) dovendosi prima procedere a studi geologici e specialistici di microzonazione di terzo livello. Ecco perché occorrerebbe delocalizzare la ricostruzione, ad esempio

Ciò al fine di ottimizzare le risorse e salvaguardare l'incolumità della popolazione. Faccio questa precisazione perché localmente anche qualche sindaco affermò,

Sul territorio, con attivisti, sindaci, comitati di cittadini, ingegneri e geologi, abbiamo creato un tavolo tecnico dal quale sono scaturite una serie di proposte emendative, la cui pertinenza e validità sono assicurate dall'osservazione sul campo e dall'ascolto delle esigenze dal basso. Quindi, si è operata un'attività normativa che ha decodificato esigenze reali e non supposte tali, con procedimento induttivo. Di fronte a un'Italia che già nei primi tre mesi del corrente anno ha registrato un lieve incremento del PIL (+0,l per cento) e delle trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato tra il 75 per cento siamo contenti, con questo provvedimento, di contribuire all'inversione di tendenza con soluzioni la cui ricaduta e i cui frutti, in termini di investimenti, incremento economico e stabilità sociale, si potranno rilevare solo tra qualche anno.

perché hanno veramente lavorato instancabilmente in queste settimane per concludere l'esame del provvedimento; sono stati veramente ottimi. Dopodiché, dopo una piccola pausa elettorale, a questo punto continua l'azione di questa Assemblea che - è ormai chiaro - incontra il favore dei cittadini, dato il risultato di domenica scorsa. Si è trattato, infatti, di un risultato ottimo per la maggioranza, con un successo che è ancora sopra al 50 per cento dopo un anno di governo. In questa cornice ci accingiamo quindi ad approvare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge cosiddetto sblocca-cantieri, ovvero di un pacchetto di misure che puntano a far ripartire il lavoro nel settore dell'edilizia e degli appalti pubblici. Le Commissioni 8a e 13a si sono riunite a lungo nelle ultime settimane per migliorare il testo di partenza e credo che sia stato fatto veramente un ottimo lavoro, un lavoro di livello, figlio anche delle numerose audizioni che negli ultimi mesi sono state svolte in entrambe le Commissioni e che ci hanno permesso di raccogliere i punti di vista di ogni attore in campo: abbiamo audito dalle associazioni di categoria ai sindacati, dai rappresentanti degli enti locali alle partecipate statali maggiormente coinvolte negli appalti pubblici. Da una parte quindi ringrazio le opposizioni per aver apportato un contributo positivo in Commissione e aver evitato di fare dell'ostruzionismo e dall'altra mi congratulo con la maggioranza per il testo che ne è uscito e che credo in queste ore sarà poi completato con gli ultimi emendamenti del Governo.

che è stata definita dalle incessanti richieste di aiuto che ci sono arrivate dalle innumerevoli associazioni del settore, messe in ginocchio da una massa immane di norme, leggi e procedure che hanno esaltato il concetto di burocrazia fino ai limiti che solamente noi italiani riusciamo a raggiungere Abbiamo quindi agito sostanzialmente su tre fronti: sul codice degli appalti e le cantierizzazioni, sulla rigenerazione urbana e sul post-terremoti. Sul codice appalti e le cantierizzazioni abbiamo operato sulla normativa vigente, mantenendo ferme le regole necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza contro chi è disonesto, ma modificando alcune norme che erano divenute vere e proprie catene per tutta quella maggioranza di onesti appaltatori e imprenditori che chiedono semplicemente di poter lavorare.

L-SP-PSd'Az)*. Per qualcuno la responsabilità coincide con il parlare solo ed esclusivamente di debito pubblico; per noi invece è irresponsabile non legiferare per la crescita e l'aumento del PIL

dall'inizio della crisi, infatti, certificano che abbiamo perso 600.000 posti di lavoro e hanno chiuso 120.000 imprese nel solo settore delle costruzioni;

Siamo dunque intervenuti dando la possibilità alle amministrazioni di appaltare i lavori in modo più snello, oltre a creare le condizioni affinché le principali opere ferme da tempo potessero essere sbloccate grazie alla nuova figura dei commissari *ad acta.* Mi si permetta un piccolo inciso, perché vale anche la pena sottolineare che un emendamento a prima firma della senatrice Saponara del nostro

Sulla rigenerazione urbana abbiamo introdotto alcune innovazioni importanti, che puntano a recuperare il patrimonio edilizio esistente e deteriorato, andando a evitare un ulteriore inutile consumo di suolo. Abbiamo puntato sulla riqualificazione e il miglioramento delle strutture esistenti in termini di sicurezza, qualità abitativa e innovazione tecnologica. Sul post-terremoti, situazioni presenti in diverse zone d'Italia negli ultimi quindici anni, abbiamo messo mano alle lacune presenti nella legge vigente e da una parte abbiamo fornito ai Comuni quegli strumenti normativi che erano indispensabili per velocizzare le costruzioni, mentre dall'altra abbiamo dato ai privati cittadini la possibilità di accesso a una serie di sgravi fiscali, per essere sollevati dall'obbligo di pagamento di tasse su beni che ormai erano inesistenti o inutilizzabili (ci sembra normale). Siamo quindi rimasti fedeli alla nostra idea che chi lavora in questo settore non può e non deve essere considerato un furbetto a prescindere, piuttosto deve essere aiutato a svolgere bene il proprio lavoro, perché noi di base crediamo che gli amministratori lavorino per il bene della propria comunità e siamo certi che i bravi imprenditori generino occupazione, rischiando spesso del loro e ottenendo sovente ben poche soddisfazioni. Sto dicendo cioè che là, a casa, dietro la parola «imprenditori» ci sono delle persone che meritano una risposta dalla politica, che è mancata per troppo tempo. *(Applausi Se poi qualcuno sbaglierà, questo dovrà pagare pesantemente il conto alla giustizia; mi sembra una cosa più che ovvia. Concludendo, signor riteniamo che questo provvedimento segni una discontinuità importante con il passato e siamo fieri, come Lega, di poter dire che abbiamo raccolto le richieste di un importantissimo settore in crisi per un possibile rilancio, trasformandole

Penso sia encomiabile l'intento, che tutti i Governi si sono posti, di sveltire il sistema degli appalti; ritengo che sia una materia delicatissima. A mio avviso, queste modifiche sostanziali e importanti sono già il nuovo codice degli appalti, perché, se fra tre o sei mesi facciamo un nuovo codice, rischiamo di cambiare di nuovo e di perdere altro tempo. Invece qui viene detto (luci)

Secondo me far partire i cantieri è importantissimo - come hanno già sottolineato altri colleghi - e risolverebbe tanti problemi. Crescerebbe il PIL, crescerebbe l'occupazione e migliorerebbe l'ambiente, perché oggi si costruiscono opere pubbliche con criteri diversi, si piantuma nelle aree libere, si evitano le code alla circolazione, aumentando la possibilità di circolare sulle strade e nelle circonvallazioni attorno alle città. Si migliorerebbe inoltre il bilancio,

aree degradate; parlo dei fondi a favore degli enti locali. Anche i fondi dell'ANAS hanno delle procedure di appalto molto lunghe; quindi sono rimasti dei residui nei bilanci degli enti locali, degli enti a ciò deputati o dello Stato.

un tecnico di un Comune fino a 5.000 abitanti, un tecnico di un Comune fra i 5.000 e i 20.000 e così, a seconda della classe demografica, un tecnico di una Provincia, un tecnico dell'Anas ingegneri, architetti, geometri e anche degli amministrativi - quelli che curano le procedure d'appalto - perché avrebbero potuto dirci dove si annidano i problemi nelle procedure di appalto. Scorrendo brevemente i testi di alcuni articoli, mi viene da dire

che comportino la sostituzione di parti strutturali delle opere, procedendo sulla base del progetto definitivo, perché si accelera un passaggio, che è quello del progetto esecutivo. Si prevede però - e questa è un'ombra - di dare una diversa definizione del progetto di fattibilità che tenga conto del minor consumo di suolo possibile - credo che questo sia implicito - e, attraverso un emendamento, del miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Io credo che questi documenti - abbiamo visto quello per la TAV - possano essere tirati da tutte le parti e quindi possano essere - per così dire - di comodo. Inoltre, del progetto di fattibilità per le opere sopra soglia bisogna redigere altri documenti - e questa è un'altra ombra studi di fattibilità ambientale e paesaggistica, la descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale. Credo che tutto questo sia già compreso nel progetto generale. C'è un articolo, che invece giudico importante, di modifica dell'articolo 31 che demanda all'ANAC l'adozione di linee guida per la definizione del compito del RUP delle funzioni e anche dell'indennità al RUP, quella

al RUP va soltanto a una persona fisica, si crea un'eccessiva disparità rispetto agli altri componenti degli uffici e ciò determina, viceversa, il blocco dei lavori. Approvo la modifica apportata all'articolo 36 in materia di contratti sotto soglia, allorché si va a stabilire, anche in difformità rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, che da 40.000 a 150.000 si possono

riguarda la norma che prevede che la stazione appaltante per i contratti sotto soglia possa procedere all'aggiudicazione di norma, sulla base del criterio del minor prezzo,

perché permette una valutazione di altri parametri; mentre quello del puro prezzo può creare problemi, perché può andare a scapito della qualità o portare contestazioni in sede di contabilità finale.

e ha generato tutta una serie di problematiche di costituzione e funzionamento. La possibilità di considerarla facoltativa sarà dunque ben accolta.

incontro a parametri di giudizio che non risentano della crisi. La modifica dell'articolo 97 in materia di offerte anormalmente basse rivede il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basandolo su un solo criterio e su una formula che non permetta l'eventuale accordo tra i partecipanti. L'articolo 4 del decreto-legge reca disposizioni in materia di commissari straordinari e mi trova assolutamente d'accordo. Un tempo, i commissari erano di norma i Presidenti delle Regioni: oggi non è più così, ma è da valutare. Quando si farà l'elenco dei commissari straordinari, prenoto l'opera Asti-Cuneo, che è il classico caso in cui possiamo inserire un'opera che sta faticando nel sistema del commissario straordinario, che ha poteri speciali nell'eventuale rielaborazione dei progetti del sistema di appalto, e via Per quanto riguarda il sistema delle opere collegate ai terremoti o ai disastri naturali,

penso che il Governo o i Presidenti di Commissione, alla luce delle osservazioni fatte e degli emendamenti presentati, possano apportare lievi modifiche costruttive e procedurali.

onorevoli colleghi, l'Italia è geologicamente molto fragile e i grandi rischi naturali - sismico, idrogeologico e vulcanico - la affliggono da Nord a Sud. La pericolosità dei fenomeni naturali e la vulnerabilità del costruito determinano rischi molto elevati, con soglie gigantesche lungo tutta la dorsale appenninica. Siamo flagellati mediamente da un terremoto distruttivo ogni quattro anni e mezzo e a ogni terremoto ci ritroviamo a fare la conta dei morti e dei danni e a intervenire in emergenza, durante il terremoto con misure di protezione civile e dopo di esso con ricostruzioni molto spesso problematiche. Sappiamo bene che solo la prevenzione può mitigare il rischio sismico, ma la politica su tale pratica è sempre stata latitante. questo Governo ha intrapreso un virtuoso percorso verso la prevenzione dei rischi naturali, unica via in grado di garantire la sicurezza del territorio e salvaguardare la vita. È arcinoto che, con la spesa imposta dalle provvisorie e rabberciate emergenze, si può investire in durevole e accurata prevenzione. Purtroppo, in assenza di prevenzione, inseguiamo i disastri. Alla gravosità della fase emergenziale segue la lentezza della ricostruzione, a causa sia delle difficoltà oggettive di ripristinare territori devastati, sia delle pessime gestioni politico-amministrative passate. In questo anno di Governo ci siamo già occupati del superamento di ritardi e inadempienze accumulatesi nelle passate ricostruzioni *post* terremoto. Qui ci occupiamo, tra l'altro, dell'accelerazione degli interventi infrastrutturali e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il capo II reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise (sismi di Montecilfone del 15 e 16 agosto del 2018, con magnitudo 4,7 e 5,1) e dell'area etnea (sisma di Zafferana etnea del 26 dicembre 2018 con magnitudo 4,8). sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili; l'assistenza alla popolazione; la ripresa economica dei territori dei Comuni colpiti dai terremoti citati. Si dispone la nomina dei commissari straordinari per la ricostruzione dei territori dei Comuni molisani e della Città metropolitana di Catania, che provvedono, attraverso specifici piani di trasformazione ed eventualmente di delocalizzazione urbana, alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica con un finanziamento di 276 milioni di euro nel prossimo quinquennio. Tra le funzioni elencate vi è la possibilità di dotare i Comuni di un piano di microzonazione sismica di terzo livello, la più approfondita possibile prevista. Sottolineo lo spirito di tali prevenzione di tali competenze: mitigare i rischi naturali e studiare la risposta sismica del sisma per un corretto adeguamento antisismico delle strutture. L'articolo 10 detta criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata differenti a seconda del danno. L'articolo 13 è dedicato alla demolizione, ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. È, inoltre, previsto un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture. riparare i guasti antichi del territorio per prevenire ulteriori gravi conseguenze nei sempre più frequenti estremi fenomeni atmosferici inaspriti dal cambiamento climatico in atto. Il capo III reca disposizioni relative agli eventi sismici del 2009 dell'Aquila, del 2016 e 2017 del Centro Italia e del 2017 dell'isola d'Ischia. L'articolo 21 prevede un contributo straordinario di 10 milioni di euro al Comune dell'Aquila per il 2019 e di altri 10 per il 2020. L'articolo 23 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 per accelerare la ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016-2017. Si dispone un aumento del contributo aggiuntivo previsto per le attività tecniche finalizzate all'analisi di risposta sismica locale, che concretamente permettono di adeguare le strutture a rischio sismico del sito di fondazione. Ulteriori disposizioni del capo III riguardano il codice della Protezione civile per esemplificare le procedure per il ristoro dei danni alle attività economiche e produttive e ai privati a seguito di eventi calamitosi. Ristoro dei danni delle calamità naturali; aiuti ai territori; ricostruzione e tutela dei beni culturali e paesaggistici; attenzione alle infrastrutture; accelerazione degli interventi; semplificazione delle norme; mitigazione del rischio sismico e idrogeologico e prevenzione sono le parole d'ordine del decreto-legge Tanto si può ancora fare per mitigare i grandi rischi naturali, a cominciare dalla conoscenza del territorio. Sono, infatti, auspicabili una maggiore copertura di stazioni sismiche a mare, studi sulle strutture sismogenetiche e modelli crostali di velocità di propagazione delle onde sismiche, per una più precisa localizzazione dei terremoti costieri e una migliore valutazione della pericolosità. È, poi, indispensabile il rifinanziamento della moderna cartografia geologica, fortemente deficitaria proprio nelle aree a maggior rischio, basilare strumento scientifico per una corretta gestione del territorio. Stiamo costruendo, tassello dopo tassello, quella necessaria sicurezza del Paese per tanto, troppo tempo negata. Il faro del bene collettivo per il MoVimento 5 Stelle è sempre luminoso.

In verità, si destrutturano le norme sulla legalità e la trasparenza. Io ascolto i colleghi sempre con molta attenzione, in primo luogo quelli del MoVimento 5 Stelle. Ma state parlando di un altro decreto-legge, non di questo. State parlando di un'altra storia, non di questo decreto-legge. Qui si destrutturano tutte le norme sulla legalità. nostro Paese è pendolare. Rileviamo che ci sono dei problemi sulla legalità e si fanno un po' di norme sulla legalità; poi scopriamo che i cantieri non vanno avanti e, quindi, si destrutturano le norme sulla legalità. Faccio solo un esempio. Noi abbiamo svolto una discussione e facciamo anche delle valutazioni comuni - come per esempio - sul tema degli incidenti nei cantieri. Sia chiaro, però, che, se aumentiamo il subappalto

in relazione al tema del subappalto e della crisi che ha attraversato l'impresa dell'edilizia, che ha prodotto imprese che di fatto non hanno struttura e sostanzialmente utilizzano manodopera. Questo è il problema dell'Italia. Quante sono le imprese vere nella gestione dell'edilizia? Ho

abbiamo una pubblica amministrazione non in grado di gestire gli appalti pubblici. Se vogliamo gestirli con serietà, bisogna assumere tecnici, ingegneri, progettisti, personale capace di occuparsi della direzione dei lavori, e di fare il RUP, che oggi non abbiamo nella pubblica amministrazione.

corruzione e aumento dei costi della pubblica amministrazione. Quante varianti si faranno? Come e chi controllerà le varianti? Come sono le stazioni appaltanti? Qual è il livello di qualificazione delle stazioni appaltanti? Sapete quante stazioni appaltanti qualificate abbiamo oggi in Italia? Lo chiedo al Governo, ai relatori. Rispondetemi nella replica: quante stazioni appaltanti qualificate abbiamo nel nostro Paese oggi?

danno alla pubblica amministrazione e alla capacità di risolvere i problemi. Presidente, noi di Fratelli d'Italia siamo in profonda sintonia con chi sostiene un grande e non più rinviabile piano di sviluppo infrastrutturale che rimetta in moto la nostra economia. Ce lo chiedono le nostre aziende, i nostri imprenditori, i nostri Comuni, i nostri territori e le categorie che abbiamo audito in Commissione.

e cioè quella di voler certificare il dramma delle nostre opere pubbliche che sono ingabbiate, mortificate, frustrate da un mostro che si chiama burocrazia. questo mostro che sconfina nei meandri della pubblica amministrazione, in realtà, incide sulla natura stessa del dirigente e del politico. Io - come credo molti in quest'Aula - ho avuto la fortuna di essere assessore ai lavori pubblici nella mia città. Devo dire che

La stessa cosa - devo dire - tocca al dirigente dello Stato italiano che di buon grado fa finta di niente, mette la testa sotto la sabbia e purtroppo

la realizzazione delle opere. Bisogna intervenire sulla burocrazia nella fase autorizzativa delle opere, eliminare quegli ingiustificabili allungamenti di tempi, di messa a bando, di valutazione di appropriazione, di firma del contratto e di pagamenti che paralizzano gli operatori economici e, quindi, i cittadini. Ho sentito gli amici della Lega condividere il problema. Noi siamo preoccupati per questo. Sono consapevole che abbiamo finalmente individuato una delle cause dei mali della nostra Nazione, ma riteniamo necessaria una sorta di di rivoluzione culturale, perché consideriamo gli appalti pubblici - i cantieri, di cui si è abbondantemente discusso - un'occasione fondamentale di sviluppo. Avete indovinato il nome - come spesso accade a questo Governo

Ecco perché noi di Fratelli d'Italia ci battiamo e ci batteremo sempre affinché quest'Assemblea possa vedere approvati provvedimenti che noi chiameremmo, più che sblocca cantieri, spazza burocrazia.

purtroppo non solo inutile, ma - io ritengo - anche dannosa. Avete di fatto deciso - lo ha detto bene il collega, senatore Errani - di smontare il codice degli appalti, nell'idea - francamente smentita dai numeri che esso sia causa dello stallo delle opere pubbliche. Non è così. L'anno scorso le opere pubbliche, i bandi e le aggiudicazioni hanno avuto un incremento netto e deciso, come dimostrato dai dati del Cresme. La tesi è quindi fallace.

consentendo persino di non far più affidamento alle centrali di committenza, che erano un primo importante passo in avanti.

Magari! L'ultima volta il regolamento ha avuto bisogno di quattro anni per essere approvato. Per tutto il tempo durante il quale il regolamento non sarà approvato rimarranno in vigore linee guida che fanno riferimento a un codice superato dal provvedimento in esame. La confusione nelle stazioni appaltanti sarà enorme e la difficoltà di affidare lavori, seguirli e farli realizzare compiutamente e correttamente sarà ancora più grande. Altro che sblocca cantieri! Vi sfido: vedremo di qui a qualche mese quante gare si sono invece bloccate.

degli elementi criminogeni e pericolosissimi sotto il profilo della trasparenza. La soglia della legalità si abbassa di tanto. Peraltro, non abbiamo neanche

con possibilità di affidare i lavori per trattativa privata, senza una vera e propria gara. Addirittura si torna al meccanismo del prezzo più basso sino alla soglia di 5,5 milioni di euro, e noi l'avevamo fissata

Si aboliscono gli albi dei direttori dei lavori e dei collaudatori nei *general contractor*. Si tratta di una cosa assolutamente folle, perché si dà così la possibilità a un *general contractor* di affidare, *intuitu personae,* incarichi (anche del valore di milioni di euro)

e, soprattutto, la distinzione tra l'impresa che realizza e il progettista terzo, rispetto tanto all'amministrazione quanto all'impresa. Al contrario, si mette di nuovo il progettista sotto le grinfie dell'impresa,

nominato un commissario: teoricamente, su tutte. Non si dice che tipo di criteri deve avere il commissario, di onorabilità e di professionalità, per svolgere il ruolo e, soprattutto, si scrive che può operare in deroga alle leggi. Gli si dà un potere enorme, questo sì criminogeno. Contro queste cose domani ci batteremo fino in fondo e speriamo davvero di essere ascoltati.

Il decreto-legge si occupa principalmente della ricostruzione del sisma che lo scorso anno ha colpito il Molise e parte della Provincia di Catania, in Sicilia. Si prevede qui la nomina di due commissari straordinari alla ricostruzione, uno per ciascuno delle due aree, scelti d'intesa con i Presidenti regionali. Si prevede lo stanziamento di una dotazione di quasi 260 milioni per cinque anni per far fronte alle spese. Per la ricostruzione privata, si prevede il riconoscimento del danno fino al 100 per cento delle spese sostenute. Si prevedono la ricostruzione pubblica di edifici pubblici, chiese, beni culturali e interventi per assicurare servizi con procedura negoziata. Si istituisce una zona franca urbana per le imprese e anche per i professionisti. Poi interveniamo anche per il sisma dell'Aquila del 2009. Al contributo di dieci milioni alla città dell'Aquila, già previsto per quest'anno, in fase emendativa ne abbiamo aggiunti altri dieci per il 2020. E si spera di approvare domani la proroga, per tutto l'anno del termine per le imprese per la comunicazione dei danni subiti e le osservazioni, in ordine al provvedimento aperto dalla Commissione dell'Unione europea per gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi. Soprattutto, in questo decreto-legge interveniamo ancora con tante misure per il terremoto del Centro-Italia del 2016 che, di fatto, è e sarà per moltissimi anni il più grande cantiere del Paese, quello della ricostruzione, che deve dare speranza

il decreto proroga termini di luglio, con il decreto per Genova di settembre e con la legge bilancio 2019, altre nuove misure sono state apportate in questo decreto, già alla sua emanazione, e altre sono state ulteriormente migliorate e incrementate in fase di conversione. È la conferma, signor Presidente, colleghi, che questa maggioranza, soprattutto la Lega e il ministro dell'interno Salvini, hanno a cuore le comunità terremotate, alle quali non è mai mancato e mai mancherà in futuro il sostegno. Ricordo che nei suddetti quattro provvedimenti abbiamo inserito moltissime misure, oltre a beneficio delle famiglie e delle imprese. Abbiamo modificato norme urbanistiche, apprezzate da quasi quarantamila professionisti che operano nell'area del cratere, tra ingegneri, geometri, architetti e geologi. Per esempio, abbiamo regolarizzato - e ci tengo a ricordarlo - le piccole difformità su edifici privati che paralizzavano gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati. Abbiamo inserito - lo ricordo - molte misure fiscali, come la proroga al 2020 della zona franca urbana, aumentando da 60 a 120 le rate della busta paga pesante, e abbiamo escluso sino al 2020 dal reddito i fabbricati inagibili ai fini del calcolo dell'ISEE, ai fini Irpef e del reddito delle società. Con questo decreto, soprattutto per il Centro-Italia, stiamo lavorando ancora in queste ultime ore e negli ultimi minuti per il cantiere più grande del Paese. Sbloccare per ricostruire: è così che la Lega intende da sempre il suo impegno nei confronti delle comunità terremotate. La Lega vuole i Comuni protagonisti nella ricostruzione e abbiamo creato le condizioni affinché i sindaci e i Comuni

Questa misura, unita a quella che prevede l'assunzione presso gli stessi Comuni di 350 dipendenti a tempo determinato, che mi auguro possa essere approvata domani, determinerà una svolta epocale nella ricostruzione. Per i Comuni, ancora, è stato previsto il ristoro dell'esenzione della tassa di pubblicità e della tassa di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali commerciali nel cratere, che quindi hanno avuto un ulteriore aiuto da parte di Governo e Parlamento. Per la ricostruzione pubblica si prevedono notevoli semplificazioni per gli affidamenti degli incarichi di progettazione: affidamenti diretti per incarichi inferiori ai 40.000 euro e per soglie superiori procedure negoziate semplificate. Per i privati, invece, abbiamo introdotto ancora un'ulteriore proroga di quattro mesi del termine per l'avvio della restituzione delle rate della busta paga pesante: in sostanza, i primi rimborsi, anziché scattare dal mese di giugno, saltano alla fine di ottobre di quest'anno. È stata estesa per il 2019 l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro

il divieto di vendita dell'immobile distrutto e inagibile già beneficiario di contributo, che di fatto impediva gli interventi di ricostruzione. Altre novità importanti sono - ad esempio - i criteri stabiliti per evitare la concentrazione di incarichi contemporanei ai professionisti nella ricostruzione privata: cosa non superflua - lo sottolineo - visto che pochi tecnici intraprendenti hanno creato veri e propri monopoli rappresentando, lì nel cratere, degli imbuti e, dunque, dei rallentamenti negli interventi. Che dire poi della norma che, rispettando il testo unico dell'ambiente, ha introdotto finalmente il limite alla presenza di amianto nelle macerie? Eviteremo finalmente il blocco delle rimozioni, accaduto moltissime volte in passato, anche per la sola presenza di una piccola quantità di questo rifiuto pericoloso. L'ultima misura introdotta che voglio sottolineare è quella che mira a scongiurare i fenomeni di spopolamento e di abbandono soprattutto nei piccoli paesi. *(Applausi i Comuni che presentano oltre il 50 per cento di immobili dichiarati inagibili e distrutti si prevede l'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili. Lasciatemi dire che nonna Peppina con la sua casetta, per la quale - lo rivendichiamo - la determinazione della Lega ha consentito il dissequestro e dunque l'uso, ha rappresentato un esempio da poter seguire e autorizzare in tutta l'area del cratere. Presidente, mi avvio a concludere, non prima di aver ringraziato per il tanto e positivo lavoro svolto i relatori Faggi e Santillo, i colleghi delle Commissioni ambiente e lavori pubblici, il vice ministro Rixi, il sottosegretario Crimi e, soprattutto, gli Uffici, che hanno sviluppato un'enorme mole di lavoro. Per le comunità terremotate resta ancora molto da fare, però siamo convinti come Lega che, continuando ad ascoltare i territori colpiti, le popolazioni,

stiamo veramente definendo sempre di più misure e strumenti per fare bene e accelerare le ricostruzioni. In occasione delle recenti elezioni europee

molte delle quali vanno a pezzi - hanno dato oltre il 40 per cento di consensi alla Lega, un dato che certifica che i cittadini e gli imprenditori colpiti dal sisma stanno apprezzando il nostro impegno, nostro impegno, decidendo di riporre ancora in questo Governo e nella Lega la loro fiducia per una rapida ricostruzione.

non sblocca cantieri» è la migliore valutazione su questo provvedimento che ho sentito in Commissione nel corso delle audizioni degli esponenti dei vari mondi economici e imprenditoriali e delle associazioni rappresentative dei nostri enti locali. Molte, anzi moltissime sono le criticità di questo testo. È evidente l'intento del Governo di mettere una pezza per frenare lo sconcerto dell'opinione pubblica e delle imprese causato dall'estemporaneità di fermare le opere pubbliche del Paese. come sempre avviene mettendoci una pezza, il risultato prodotto non è risolutivo e ottimale e la proposta risulta parziale, insufficiente e in molte parti sbagliata. alcune considerazioni. Innanzitutto, va rilevato che tra le pieghe del decreto-legge, che dovrebbe essere un provvedimento urgente, sono previsti almeno 15 decreti e provvedimenti attuativi che deve adottare il Governo, ma non solo. Per Per l'adozione del Regolamento unico, per esempio, che sostituirà le linee-guida ANAC e i decreti attuativi del codice degli appalti, la scadenza è fissata al 19 ottobre. I tempi, quindi, non saranno quelli di norme immediatamente operative, come richiederebbe lo stallo delle opere pubbliche. Stesso discorso vale per i commissari straordinari, che dovrebbero occuparsi degli interventi infrastrutturali prioritari, per nominare i quali sono necessari uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, senza un termine perentorio, per cui campa cavallo. commissari straordinari per interventi sulla rete viaria della Regione Sicilia, per la ricostruzione nella provincia di Campobasso e per i 30 Comuni dell'area metropolitana di Catania,

(quarant'anni), Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e ricordo l'attenzione alle strade di Spoleto, che è il capofila tra i Comuni del cratere dell'Umbria. Con gli stessi decreti sono previsti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso per i commissari straordinari. Quindi, le misure principali di questo decreto-legge richiedono ulteriori norme attuative che non sono certo di brevissimo periodo. In buona sostanza, sono pochi i cantieri che riusciranno a essere sbloccati entro la fine di quest'anno; quindi, l'impatto di questo decreto-legge sulla crescita economica del 2019 sarà irrisorio, se non nullo. Molto preoccupante è il ritorno al sistema del massimo ribasso, che rischia di produrre una presunta accelerazione della realizzazione delle opere, che avverrebbe, però, solo nel momento dell'affidamento, con rischi evidenti, invece, per la fase realizzativa, che è quella più importante, derivanti da un minore contenimento degli azzardi in fase di offerta. Il prezzo deve essere allineato a riconoscimenti, referenze e certificazioni che il professionista ha in possesso. Basta fare sempre sconti esagerati e fare la guerra dei poveri. Molto evidenti sono i rischi anche per la qualità dell'occupazione. Nello specifico, negli appalti sotto-soglia è definito nel minor prezzo il criterio da utilizzare in via preferenziale, seppur corretto con il metodo di esclusione automatica dell'offerta anomala. Penso, per esempio, al personale che si occupa di sicurezza: non può essere pagato al ribasso. La revisione della disciplina dell'esclusione automatica delle offerte anomale è inadeguata all'obiettivo (di contenimento dell'eccesso di ribasso), e potrebbe favorire - ecco il rischio - il ritorno agli accordi di cartello, visto che manca un efficiente meccanismo anti turbativa. Per fortuna, anzi, grazie all'accoglimento di un nostro emendamento, è stata rivista la disciplina delle clausole di esclusione che prevedeva la possibilità

il sistema di incentivi normativi (e fiscali nel decreto-legge crescita) per innescare operazioni di rigenerazione urbana

Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha annunciato l'arrivo di un primo emendamento - lo stiamo aspettando - per dare a un commissario il compito di mettere in campo i progetti di messa in sicurezza idrica del Gran Sasso. La via dell'emendamento per accelerare singole opere o piani è, però, molto rischiosa perché può scatenare una corsa a inceppare il decreto-legge di norme *ad hoc* anziché fare un accordo, presto e bene, sulle opere e sui piani da sbloccare con un decreto di Palazzo Chigi. Senza questo passaggio-chiave che avvii veramente la stagione dei commissari, l'ambizione di riavviare in tempi rapidi la spesa resterà tale. Senza contare, poi, il rischio *boomerang* di una nuova frenata dei bandi a causa della necessità delle stazioni appaltanti di adeguare documenti e procedure alla raffica di novità in arrivo. Il decreto-legge nel suo insieme mi sembra, dunque, contorto non fruibile nell'immediato. Si rischia di complicare lo stato di fatto, riguarda poco l'aspetto ambientale e viene quasi tutto concentrato nelle Regioni del Sud, ma ricordo che i grandi sismi sono avvenuti anche in Regioni del Nord, come il Friuli, che non viene minimamente nominato.

Consiglio di porre veramente attenzione alla prevenzione, investendo risorse ora per risparmiare in futuro, e non risparmiare soltanto denaro, ma molto spesso vite umane. Il nostro territorio è fragile. Infatti, come si fa a parlare di sismologia, interventi e altro se non abbiamo ancora ricoperto l'Italia con le carte geologiche, con i progetti Cargo che ci permettono di sapere e di prevenire, con una mappatura geologica complessiva, prima di prevedere nuove opere pubbliche o edilizie? Altrimenti richiamo di costruire sull'argilla. È quindi necessario fare da subito le carte geologiche. Sarebbe come costruire un grattacielo senza il progetto. Nello sblocca cantieri vi è ancora troppo potere all'ANAC, ma chi seguirà lo specificherà. Le amministrazioni locali, che sono le più preoccupate, confermano il disorientamento dei funzionari pubblici locali: per i Comuni sono troppe le variabili da considerare, gli adempimenti da effettuare e gli atti da emanare successivamente all'adozione del nuovo codice, con confusione normativa e contraddittorietà rispetto alla giurisprudenza in materia, con linee guida talvolta considerate poco chiare. Sono assolutamente condivisibili molti passaggi della Corte dei conti che abbiamo ascoltato, in cui si evidenzia la sussistenza di diverse problematiche ricorrenti che possono raggrupparsi in due grandi questioni, una delle quali è la difficoltà da parte delle stazioni appaltanti di applicare correttamente la normativa in tema in tema di individuazione del contraente, con frequente ricorso all'affidamento diretto, anche al di fuori dei casi consentiti dalla legge e di utilizzo non conforme del codice dell'istituto dell'affidamento *in house,* ovvero del ricorso alla proroga dei contratti preesistenti. Per questo tale situazione rende indifferibile un programma di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane, dei tecnici interni alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti. Molti piccoli Comuni, infatti, non hanno queste professionalità. Ne consegue dunque la necessità di procedere all'aggregazione delle stazioni appaltanti, che sono attualmente oltre 32.000, e di accrescerne dimensione e competenza.

riscrivendo da capo 13 provvedimenti del vecchio codice; totale assenza di norme per semplificare la *via crucis* delle procedure; tempi lunghi per nominare i commissari; il rischio del caos normativo. In conclusione, mancano le parole-chiave con cui il provvedimento era partito: urgenza, sblocco dei cantieri fermi, commissari subito, utilizzo dei 150 miliardi di risorse già stanziate e mai partite. Questo ennesimo provvedimento dal titolo evocativo e accattivante in realtà è un altro atto che, all'interno di una scatola infiocchettata, contiene una serie di oggettini accessori che non risolveranno i problemi infrastrutturali ed ambientali del Paese.

il decreto-legge sblocca-cantieri affronta una delle più importanti emergenze che questo Governo ha dovuto trattare da quando si è insediato: il fatto che molte risorse pubbliche, decine di miliardi di euro, non vengano spese a causa della complessità delle norme, dell'interpretabilità delle stesse e dei contenziosi che si generano. Ciò comporta forti rallentamenti per la realizzazione degli appalti pubblici, il blocco di ingenti risorse già stanziate che potrebbero essere iniettate nell'economia reale, il proliferare di contenziosi giudiziari, ma soprattutto la privazione, per i cittadini, di servizi pubblici deliberati dalle varie amministrazioni. Il mercato degli appalti pubblici, secondo le ultime stime della Commissione europea, vale oggi in media in Europa circa 2.000 miliardi di euro l'anno e solo in Italia nel 2017 circa 139 miliardi all'anno per quel che riguarda gli affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000 euro. Ricordiamo però anche che una ricerca dell'università Tor Vergata di qualche anno fa mostra come gli sprechi nel settore degli appalti sono pari a circa 30 miliardi di euro del PIL), di cui il 13 per cento è dovuto alla corruzione e l'87 per cento all'incapacità e all'incompetenza degli uffici tecnici e degli amministratori.

Questo lavoro, sintetizzato dai relatori Santillo e Faggi, insieme a quello del sottosegretario Vito Crimi, che ringrazio, sono stati fondamentali nella redazione del decreto-legge. Entrando nel merito del dispositivo normativo, vari articoli si occupano di come semplificare e ridurre l'interpretabilità della normativa specifica in materia di appalti pubblici. però concentrare il mio intervento sulla seconda parte del testo, quella relativa alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici. Io sono marchigiano e la Regione Marche è quella in cui vivo e dove ho svolto per decenni la mia attività di geologo e di ricercatore universitario. È anche una delle Regioni del Centro Italia che ha subito gli effetti più devastanti dei sismi del 2016 e del 2017. Il precedente Esecutivo aveva già legiferato con diversi decreti, a cui ne sono seguiti altri, emanati dall'attuale Governo, che, nel cambiare passo per velocizzare la ricostruzione, hanno di fatto semplificato e sanato alcune criticità (vedansi per esempio le difformità edilizie). Ora, con questo nuovo decreto-legge, si vanno ad aggiungere ulteriori misure, che porteranno a un'ulteriore sburocratizzazione. Oltre a ciò, sono stati inseriti nuovi finanziamenti per far fronte alle richieste di accelerazione della ricostruzione, riguardanti sia l'assunzione di personale che il potenziamento della struttura preposta a esaminare le richieste di contributi. Altre risorse sono destinate a compensare le maggiori spese e le minori entrate dei Comuni, incluso quello dell'Aquila, colpito dalla crisi sismica del 2007 e ancora in uno stato veramente arretrato di ricostruzione. Sono destinati maggiori contributi per le esigenze degli uffici tecnici dei settori locali e della scuola dell'obbligo, inclusi asili nido, viabilità e verde pubblico. Si è previsto inoltre, sempre in virtù di una netta accelerazione della ricostruzione, di dare la possibilità ai Comuni interessati di gestire la procedura relativa agli edifici interessati da danni lievi, d'intesa con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Sui danni lievi però - scusatemi se esco un po' dall'aspetto tecnico del decreto-legge - mi è necessario ricordare quante risorse pubbliche sono state sperperate per puntellare gli edifici con danni lievi, invece di dare fin da subito la possibilità ai privati di agire direttamente con la riparazione dei propri edifici, per poi rendicontare la spesa. Viene il dubbio che queste politiche scellerate scellerate non siano state guidate da interessi pubblici; personalmente credo che sia necessaria l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per verificare come siano stati spesi i miliardi di euro destinati all'area del sisma, sia per i puntellamenti, sia anche per realizzazione delle aree SAE. Si ricorda, a chi non ne fosse a conoscenza, che su alcuni aspetti della ricostruzione sono aperte procedure giudiziali. Per la ricostruzione pubblica, purtroppo ferma al palo per le scelte scellerate ed errate di chi ci ha preceduto, con questo decreto-legge viene estesa la possibilità di affidamenti di servizi tecnici, inclusa l'elaborazione della pianificazione urbanistica e i servizi sotto soglia, previa consultazione di dieci professionisti iscritti all'albo speciale del commissario. I servizi possono inoltre essere affidati con il criterio del minor prezzo e non del massimo ribasso, come molti hanno paventato. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Il minor prezzo, facilmente calcolabile tramite un algoritmo, impedisce che si facciano ribassi esagerati, che poi si ripercuotono sulla qualità dei materiali e sulla professionalità del personale utilizzato. Di estrema importanza è l'aumento delle spese riconosciute dal commissario ai professionisti per indagini e prestazioni specialistiche, come la risposta sismica locale (che sinora non era neppure contemplata), le analisi geologiche, le relazioni ambientali e paesaggistiche. Queste analisi permettono di elevare enormemente le soglie di sicurezza e dunque di affrontare eventuali sismi futuri con maggior serenità. Sono inoltre ridefinite le soglie di pericolosità delle macerie che contengono amianto, permettendo di trasportare in discarica ammassi di rocce e terre con percentuali veramente risibili di amianto. È stata inoltre prevista una compensazione delle minori entrate nei Comuni a seguito dell'esenzione delle imposte comunali sulla pubblicità e del canone di autorizzazione per l'occupazione di aree pubbliche. Un articolo riguarda la semplificazione delle procedure per il ristoro dei danni subiti da attività economiche che sono state portate fuori Regione. È una misura che riguarda i settori a cavallo fra le quattro Regioni interessate dal sisma. La rapida elargizione del contributo permetterà di riprendere l'attività, talora a poca distanza dal luogo originale danneggiato, garantendo che il territorio non si spopoli ed evitando uno dei principali problemi dell'area sismica. Una delle disposizioni più salienti del decreto consiste nelle procedure di attivazione del sistema di IT-*alert,* che nessuno ha menzionato. Le tecnologie attuali permettono di inviare in tempo reale messaggi di allerta in caso di calamità. È una norma che il Paese attendeva da tempo e che dovrà progressivamente essere estesa a tutte le Regioni. In pratica, durante un evento, l'ufficio preposto lancia un allarme avvertendo chi è munito dei più semplici recettori, come un semplice telefonino, di che aree o strade evitare e di come comportarsi per fronteggiare la calamità e l'emergenza. Il Governo del cambiamento con questo decreto porta un contributo sostanziale non solo all'accelerazione dei processi di ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, ma inizia un percorso virtuoso per affrontare in modo funzionale e immediato le emergenze. Vogliamo che i nostri stupendi territori colpiti duramente dalle calamità naturali tornino il prima possibile alla normalità, attraverso la ricostituzione delle comunità locali, la crescita economica e la fruibilità delle aree. Noi lavoreremo incessantemente per questo.

Signor Presidente, cercherò di essere rapidissimo. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che questo provvedimento non è risolutivo di tutto il codice dei contratti perché, come ricorderanno, all'interno all'interno della nostra Commissione abbiamo incardinato il disegno di legge delega al Governo per il riordino di tutta la materia; invece, da quanto emerso durante la discussione, sembra quasi che l'intento fosse di riuscire a risolvere le problematiche dei contratti in Italia con questo provvedimento, ma così non è. Il provvedimento è un cosiddetto sblocca cantieri, perché per noi per colpire il cancro vero degli appalti in questo Paese bisognava colpire le procedure di aggiudicazione ed è così che abbiamo voluto intervenire cambiando paradigma e, anziché preferire l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti sotto soglia, passiamo all'offerta aperta con procedura al minor prezzo. Ricordo che questa è una procedura trasparente e nulla c'entra con la possibilità né che vi siano più incidenti sui luoghi di lavoro, né che ci siano lavoratori in nero. Lo stesso dicasi per il fatto che il PD legava prima la materia alla percentuale di subappalto. Voglio ricordare che ci sono alcune infrazioni segnalate dall'Unione europea come l'obbligo dell'Italia di andare verso il 100 per cento del subappalto, non ce la sentiamo, abbiamo incrementato fino al 40. Posso anche dire che anche la volontà di fare in modo che il concorrente non possa essere subappaltatore è indicata dall'Europa, ma sappiamo bene come va nel nostro Paese il lavoro e quindi per noi quella può essere una via per accordi di cartello che va assolutamente vietata, in quanto dietro vi si possono annidare le mafie. In conclusione, vorrei ricordare alla senatrice Gallone che il terremoto che c'è stato in Irpinia ha lasciato non solo dei morti, ma gravi ferite sul territorio, quindi la Lioni-Grottaminarda si innesta in uno di questi percorsi, per recuperare le infrastrutture e per far sì che i cittadini possano spostarsi da una Regione all'altra.

Concludo dicendo che in Commissione abbiamo fatto un buon lavoro, alcuni emendamenti sono stati collegiali, come ad esempio quello volto a rimuovere il massimo del 30 per cento dell'offerta economica all'interno dell'offerta economicamente più vantaggiosa e soprattutto negli articoli dal 6 al 20, finalmente in questo Paese si è intervenuti in aiuto di quelle popolazioni colpite da eventi sismici fino ad oggi forse dimenticati.

riferita al sisma, sia la parte riferita alla questione del codice degli appalti. Vorrei anche ricordare una cosa importante: il codice degli appalti per cento anni è stato regolato da un regio decreto del 1985.

vede, senatore Grasso, l'ho sempre seguita con grande attenzione come magistrato, ma non penso sia una norma a poter

l'intervento con la situazione emergenziale. Chi è stato con la Protezione civile e i Vigili del fuoco semplicemente in visita nei luoghi colpiti dal sisma sa che spesso, prima dell'avvio dei lavori e di vedere qualcosa, la terra deve assestarsi perché la natura è difficile da controllare. Ritengo si tratti di un buon provvedimento, che non abbia la pretesa di risolvere tutto, ma abbia la condizione, la volontà, la forza e, soprattutto, la determinazione di continuare in quel percorso normativo, che dura che dura da più di cento anni e che ci vede ancora qui anche se siamo quasi nel 2020, per cercare di venire incontro alle diverse esigenze che ciascuno di noi porta e che, nelle loro differenze, devono comunque essere ascoltate. Signor Presidente, abbiamo seguito il dibattito e i tanti interventi. Ringrazio i colleghi che hanno approfondito alcuni aspetti,

Vi è una narrazione che non è corrispondente alla realtà. C'è chi sostiene che il codice degli appalti in vigore ha sostanzialmente rallentato il Paese e bloccato le opere più importanti. In realtà, guardando i dati, così come anche c'è stato esposto sia nell'indagine conoscitiva che nelle audizioni successive, il codice degli appalti ha ridotto i fenomeni corruttivi. L'Italia è cresciuta nella speciale classifica dei Paesi dove c'è meno corruzione e gli affidamenti di incarichi solo nel 2018 sono cresciuti del 30 per cento.

la revisione del codice degli appalti assolutamente non è corrispondente alla realtà. Certo, ci sono dei problemi e abbiamo cercato di affrontarli con le nostre proposte e i nostri emendamenti. Ad esempio, la vostra proposta di revisione del codice degli appalti, pomposamente chiamata «sblocca cantieri», non affronta i nodi che tantissimi amministratori di tutte le parti politiche hanno più volte sollevato e non sono le offerte economicamente più vantaggiose. Quindi, non erano le linee guida o l'oppressione da parte dell'Autorità anticorruzione; non erano le procedure negoziali o le soglie. Era ben altro. Erano i mancati finanziamenti. Se penso al taglio Anas, alle opere statali affidate all'Anas per 1,8 miliardi di euro, che sposta in avanti decine e decine di cantieri in giro per il nostro Paese, si capisce bene qual è il problema; altro che lo sblocca cantieri! Penso pure alle analisi costi-benefici (che stanno rallentando, se non bloccando alcune opere strategiche nel nostro Paese) e alla pletora delle centrali di committenza, con un Paese che fa fatica rispetto alle modifiche. Lo diceva poco fa anche il presidente Coltorti.

Non c'è nulla di questo nella proposta fatta con il decreto-legge. Anzi, viene applicato il minor prezzo, il prezzo più favorevole, il ribasso, chiamatelo come volete. Sappiamo bene che cosa ha comportato in passato: salari più bassi, cannibalismo tra le imprese, meno qualità, meno sicurezza sui cantieri (con quello che potrebbe succedere). Oppure l'eliminazione del divieto di subappalto alle ditte che hanno partecipato alla gara: ma che cosa significa questo se non un accordo, un cartello tra le imprese che partecipano all'appalto per poi spartirsi l'appalto medesimo? Riduzione del ruolo dell'ANAC e affidamento ad un regolamento che sarà redatto dal Governo entro centottanta giorni: io immagino che di questo regolamento faranno parte le linee guida ANAC. Ma se le linee guida ANAC sono state un problema perché bloccavano gli appalti in questo Paese, come faremo a superarle se poi le porterete anche nel futuro regolamento? Quindi un dibattito, quasi un esercizio retorico, quello che ci viene presentato. Elevare la soglia Elevare la soglia a 150.000 per gli affidamenti diretti sappiamo bene cosa significa. Vogliamo tornare a quel sistema? Era colpa dell'ANAC o era il Paese che andava in una determinata direzione? E nel momento in cui aumentiamo le stazioni appaltanti, si polverizzano o no le esperienze, anziché centralizzarle, almeno a livello provinciale, non dico a livello di Comune capoluogo? Quindi intravedo in futuro l'aumento dei fenomeni corruttivi. Su questo noi siamo intervenuti con numerose proposte; vedremo nel dibattito parlamentare. Signor Presidente, chiudo con una chiosa finale sui commissari. Noi abbiamo ritenuto che i poteri assoluti che darete ai commissari di derogare numerose procedure sia un fatto negativo. Ma almeno ne valga la pena. Se proprio volete nominare dei commissari straordinari, fatelo *in primis* per le opere strategiche sulle quali finora avete dimostrato titubanza, se non addirittura volontà di bloccarle. Nominate allora entro pochi giorni i commissari per le alte velocità Brescia-Padova, Verona-Brennero e Terzo valico, ad esempio. Non voglio osare citare la Torino-Lione sulla quali ci sono contrarsi all'interno del Governo. Facciamo in modo che vi sia effettivamente un ritorno,

Avevamo fatto delle sollecitazioni con spirito costruttivo e ci è stato riconosciuto, l'ho detto anche prima. Non essendoci stata almeno nel dibattito - poi nel voto non sappiamo, visto che molte cose sono cambiate e basta vedere il tenore degli emendamenti presentati

Presidente, non è la prima volta che si parla di commissari straordinari. Oggettivamente, già nel 1997 il Governo Prodi intervenne attraverso la prefigurazione, la costituzione e l'individuazione di questa figura. Ma era una questione del tutto diversa, perché prevedeva l'istituzionalizzazione dei commissari straordinari per opere già previste, finanziate e bloccate.

non si riescono a realizzare, si faccia il commissario straordinario. Ed erano previsti peraltro per opere di grande valenza strategica per il Paese. Qui invece, e il dibattito di oggi non ha scalfito questa evidenza, non stiamo parlando di queste opere per due motivi fondamentali, il primo dei quali è lapalissiano: voi definite la figura di commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ma quali sono

il relatore, di opere fondamentali come, appunto, la Brescia-Padova o la Verona-Brennero. Bisogna definire un elenco.

Cittadini, territori e sindaci aspettano di fare quelle opere ed è in corso un indecente balletto con Anas e RFI, per cui queste strutture pubbliche non sanno più cosa fare e noi non siamo nemmeno nelle condizioni di sapere quali siano le intenzioni del Governo. Allora altro che commissario a prescindere, non si sa su cosa: si definisca cosa si vuole fare e dove servono i commissari e noi appoggeremo questa linea, se le opere sono davvero importanti. Si chiuda definitivamente il balletto sui contratti di servizio e si abbia la capacità di decidere.

perché ci sono varie ipotesi. Di certo si va dalle 30.000 alle 40.000. È possibile, in un Paese come il nostro, non lavorare sulla razionalizzazione e sull'aumento qualitativo di queste centrali d'appalto? Questo provvedimento, lo ripetiamo, non fa nulla. Tralascio, perché ne ho già parlato prima,

emendamento definisce che i commissari devono operare non solamente per la delocalizzazione ma anzi, prioritariamente, per per la riparazione e la ricostruzione *in loco*, perché salvaguardare il luogo dove le comunità sono state colpite e quindi la riabitazione di quei luoghi è fondamentale e di questo vi diamo atto. Ovviamente, però, rimangono tutte le zone d'ombra di cui abbiamo parlato prima e la questione fondamentale è che i Comuni, siccome sono spesso di piccole dimensioni, non hanno la competenza ma soprattutto non hanno le risorse umane nemmeno per gestire l'ordinaria amministrazione, immaginiamoci per gestire la straordinaria amministrazione, come in questo caso. Dunque noi insistiamo e ripresenteremo gli emendamenti che vanno in questa direzione.

devo dire con toni pacati e collaborazione, cercando di trovare le soluzioni. Ancora ne abbiamo di lavoro da fare, in Aula, visto che tante cose devono essere affrontate. Una cosa che mi sento di dire è che il provvedimento, nei primi cinque articoli,

del 2016, perché contengono norme di semplificazione che possono applicarsi automaticamente, in quanto introdotte nel codice degli appalti, per la ricostruzione pubblica a seguito del terremoto del Centro Italia.

aggiunge semplificazione, portando qualche elemento in più; porterà personale in più, porterà modelli diversi di elaborazione delle domande di contributo e semplificazioni.

definito, studiato e scritto dovrebbe semplicemente prenderne atto - ha fallito. Ripeto, quel modello è fallito. Questo è il motivo per cui sull'area etnea e sul Molise applichiamo un modello diverso, che mette al centro i Comuni

annullando completamente l'attuale modello, anche di *governance*, del sisma del Centro Italia, in quanto significherebbe ricominciare da zero e purtroppo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo

scegliere modalità di gestione delle istruttorie più vicine ai cittadini, che possano essere più dirette e facilmente verificabili. Infatti, oggi il grosso problema dei cittadini è che quando vogliono sapere delle proprie istanze e dell'*iter* che stanno seguendo, devono di fatto seguire un percorso a ritroso, fino a risalire a uffici sempre più lontani. Questo è il Questo è il modello che ha fallito. Rimettiamo allora al centro i Comuni. In questo momento noi rimettiamo al centro i Comuni del Centro Italia, senza imporre nulla e lasciando la facoltà di iniziare questo percorso, che sperimenteremo perché potrà solo portare qualcosa in più. Magari altri Comuni, che inizialmente non decideranno di seguire questo percorso, si allineeranno in poco tempo. Probabilmente; riusciremo anche a decongestionare gli USR, che potranno occuparsi della ricostruzione pesante, quella un po' più complessa e per la quale serve grande competenza, e di quella pubblica, che è quella ancora più problematica

Comuni: la fase iniziale più complessa, quella della progettazione dei piani urbanistici e quant'altro, era soggetta a un determinato *iter*, ma questo già prima dello sblocca cantieri era semplificato per tutto il resto d'Italia.

da accogliere perché porteranno ulteriori elementi innovativi nel processo di ricostruzione. Ringrazio nuovamente tutti. *(Applausi

a prenotarmi. Ieri, appunto, ricorreva il 45° anniversario della strage di piazza della Loggia, dove una bomba durante un comizio provocò la morte di otto cittadini innocenti e indifesi e il ferimento di altri cento. Da quel giorno vennero messi in atto ogni genere di interventi, falsificazioni, silenzi, menzogne e depistaggi, anche da parte di settori deviati dello Stato, dei servizi segreti, tutti tesi ad allontanare la possibilità di accertare la verità. Ma, ciononostante, dopo quarantatré anni dalla strage e dopo tre processi una sentenza definitiva ha riconosciuto la penale responsabilità della strage in capo a Carlo Maria Maggi e a Maurizio Tramonte, militanti del neofascismo veneto. Il primo era capo locale di Ordine Nuovo e il secondo, oltre ad essere militante della stessa organizzazione, era un informatore dei servizi segreti, celato sotto lo pseudonimo Tritone.

dei servizi segreti, ispirò una informativa all'allora SID (il Servizio informazioni difesa, cioè il servizio segreto militare), che reca la data del luglio 1974, in cui si specificava che nei mesi precedenti si erano tenute alcune riunioni di Ordine Nuovo (organizzazione neofascista ufficialmente disciolta l'anno precedente) durante le quali si era deciso di riprendere clandestinamente le attività eversive. In una di queste riunioni, tenutasi tre giorni prima Carlo Maria Maggi aveva affermato che occorreva organizzare un grande attentato e che era necessario proseguire nel solco della strategia stragista iniziata il 12 dicembre 1969 in piazza Fontana (strage anch'essa maturata negli ambienti del neofascismo veneto). L'obiettivo era incutere nella popolazione paura, caos, terrore e, quindi, creare le basi per lo scoppio di un vero e proprio conflitto nazionale che poteva aver fine solo con misure limitative della libertà e con uno scontro armato: questo, ovviamente, nelle intenzioni degli eversori. Rileggere Rileggere la sentenza di condanna sulla strage di piazza della Loggia è riaprire una ferita mai rimarginata. Dalle carte emerge che i servizi segreti e il generale Gianadelio Maletti sapevano perfettamente che cosa stava accadendo proprio in quei momenti e che cosa stavano organizzando i terroristi neofascisti, ma non li fermarono in alcun modo, né informarono i magistrati dopo la strage. Nella sentenza è scritto a caratteri cubitali che i colpevoli sono Maggi e Tramonte, ma che, leggo testualmente: «altri, parimenti responsabili, hanno lasciato questo mondo o anche solo questo Paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la malavita anche istituzionale all'epoca delle bombe». Questo fa capire - e mi avvio a concludere - il quadro complessivo di quegli anni, in cui in Italia fu combattuta una guerra non dichiarata, che alcuni a bassa intensità: da una parte, c'erano gruppi paramilitari pervasi da una folle ideologia e assetati di sangue (che, come detto, potevano utilizzare inconfessabili sponde istituzionali e contare su indicibili accordi internazionali) e, dall'altra, c'erano cittadini innocenti e inermi.